del codice penale (sequestro di persona aggravato), trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania il 23 gennaio 2019».

Signor Presidente, la questione che stiamo discutendo oggi è un precedente inquietante. Per la prima volta un tribunale dei Ministri chiede al Parlamento l'autorizzazione a processare un Ministro dell'interno che, abusando dei suoi poteri e con l'aggravante di essere un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ha privato della libertà 177 persone, alcune delle quali di minore età, e violato deliberatamente norme nazionali e convenzioni internazionali. Non era mai accaduto. Un Ministro esercita le sue funzioni giurando sulla Costituzione, giurando di essere fedele alla Costituzione e alle sue leggi, non su un contratto di Governo e, nell'esercizio delle sue funzioni, non può fare quello che vuole. Non c'è licenza di andare oltre la legge.

a tutti gli effetti, quindi una nave militare, che fa parte della Marina militare italiana attraverso il suo corpo specifico della Guardia costiera. È a tutti gli effetti su suolo italiano ed è una nave militare italiana.

è costretta per giorni e giorni a rimanere al largo, non potendo attraccare in porto. Una nave della Guardia costiera capitanata da ufficiali della Marina militare della Guardia costiera in situazione di difficoltà, perché sono persone provate, che hanno paura perché comunque può essere difficile mantenere l'ordine pubblico, perché c'è una situazione anche sanitaria che può essere complicata. Tutto questo per giorni e giorni: dirette TV, grande copertura mediatica. Comincia un'umiliante ricerca tra i vari Paesi europei invitandoli a prendersi qualche decina di migranti. Finalmente la nave può rientrare in porto. Ma perché? Perché su questo caso, sul caso di ieri - che poi si è concluso della nave Mare Jonio, sulla questione della Sea Watch c'è questo bisogno di tenere fuori dai porti decine di persone disperate? persone disperate? Questa copertura mediatica serve a far vedere che siamo robusti, che abbiamo i muscoli tesi e mostriamo la faccia cattiva rispetto a persone che in quel momento sono disperate. Stiamo parlando di alcune decine di persone, e questo serve perché si vuole dare la dimostrazione di avere risolto i problemi quando in realtà i problemi della gestione dell'immigrazione sono ancora tutti sul piatto. Ma andiamo avanti. Dopo questa copertura mediatica, arriva l'avviso di garanzia al ministro Salvini; se non ricordo male, in una diretta Facebook il Ministro lo espone e dice

Cita la sicurezza nazionale. Vedete, colleghi, la sicurezza nazionale è un tema importante. Quando si parla di sicurezza nazionale si tratta una questione di estrema importanza che riguarda certamente anche i compiti del Ministro dell'interno e riguarda molto le funzioni del Ministro della difesa. visto che ho ricoperto *pro tempore* l'incarico di Ministro della difesa, mi chiedo quale sicurezza nazionale fosse in gioco di fronte a 177 migranti salvati dalla Guardia costiera italiana. Dopo la diretta Facebook, però, un'importante ministro di questo Governo, nonché eminente avvocato, l'avvocato Bongiorno, spiega al ministro Salvini che in realtà i capi di imputazione non sono così leggeri: si parla di sequestro di persona e quindi il processo può essere complicato. Ecco che allora, immediatamente, non ci sono più dirette Facebook; non si sventolano più gli avvisi di garanzia c'è una chiamata a corresponsabilità degli altri esponenti di Governo: "Non sono solo io, ci sono il ministro Toninelli, il presidente Conte, il *vicepremier* Di Maio".

Del diritto? Delle leggi? Della giurisprudenza? Di che cosa? No. Semplicemente del fatto che loro - dicono - agiscono nel nome di 60 milioni di italiani; questo viene ripetuto come un *mantra* (non si capisce bene perché tutti gli italiani debbano riconoscersi in questo Governo): l'agire in nome del popolo italiano. Ecco che assistiamo a una di quelle giravolte su questi temi che recentemente si stanno susseguendo da parte del MoVimento 5 Stelle. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, anche se arrivava un avviso di garanzia a chiunque avesse responsabilità politica - degli altri partiti - invocava immediatamente le dimissioni. Bastava l'avviso di garanzia.

dimostrando che il collante del Governo, o meglio della poltrona su cui si sta seduti quando si sta al Governo, diventa più forte di quella che era una bandiera quasi identitaria, giustizialista, che io non condivido ma che in precedenza era sempre stata agitata. agitata. Ministro Salvini, lei ha citato anche l'articolo 52 la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino. Lei ha citato questo articolo così importante, che sta nel cuore non solo dei cittadini, ma di tutti i corpi dello Stato che devono difendere la Patria, per crearsi un salvacondotto rispetto al fatto che veniva richiesto di poter procedere nei suoi confronti per verificare la sua azione. E lo ha citato - ripeto - di fronte a 177 persone stremate che sarebbero state un pericolo per il nostro Paese.

chi arriva senza essere invitato, a chi arriva fuori dalle regole. Però, il fenomeno è talmente epocale e talmente complicato che che una sceneggiata mediatica come quella che abbiamo visto con la Diciotti, ma anche con la Sea Watch e poi più recentemente, non serve a risolvere il problema, perché dall'altro lato ci sono dei fallimenti; ci sono migliaia di sbarchi fantasma, di cui lei non parla;

Questo precedente in realtà è un grave *vulnus* per la nostra democrazia. Io dico a tutti coloro che sono in quest'Aula, di qualsiasi parte politica siano, qui non si tratta di condannare, perché non è nostro compito; si tratta di mettere i Ministri nelle condizioni di essere, come tutti, uguali davanti alla legge. Esistono norme, c'è un tribunale dei Ministri. Questa autorizzazione a procedere deve essere data.

perché a me sembra che la questione sia abbastanza semplice. Anche se in questa discussione forse non è ancora chiaro che oggi noi non discutiamo della politica sull'immigrazione del Governo: politica che io non condivido, ma che è pienamente legittima. Oggi non discutiamo della responsabilità collegiale del Governo, elemento che

elemento importante e fondamentale; ma non c'entra niente il garantismo. Noi dobbiamo rispondere a due quesiti sostanziali: l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e l'interesse pubblico preminente. Ieri, il senatore Pillon ha detto che l'interesse pubblico preminente era ed è rintracciabile in relazione alla legge sull'immigrazione, perché non tutti possono entrare indiscriminatamente nel nostro Paese. quelle 177 persone sono sulla nave Diciotti (nave militare dello Stato italiano), sono sul suolo italiano. Quindi quell'argomento non c'è. Il tema è questo: noi dobbiamo rispondere se ci sono l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e l'interesse pubblico preminente. La risposta è che Vorrei evidenziare, rispetto alla relazione di maggioranza, un punto: ho trovato singolare il fatto che l'amministrazione non funzioni più per atti,

Non ho trovato risposte sul perché il POS sia arrivato così in ritardo, eppure era una decisione che era stata assunta. Non si riesce a comprendere, in sostanza, quali sono le argomentazioni. C'era un problema per la sicurezza del nostro Paese? Credo che nessuno possa affermare questo. Si può affermare che politicamente si riteneva e si ritiene che gli sbarchi debbano essere fermati, ma questa è un'altra questione. Io vorrei che si ragionasse su un punto. Tralascio il fatto che il vice Presidente avesse dichiarato con molta

Il problema che a me interessa è sostanzialmente quello che in modo molto puntuale il senatore Grasso, nella relazione di minoranza, ha individuato: è il precedente che noi qui rischiamo di aprire. Vorrei che su questo si ragionasse. Io so bene qual è la ragione politica per la quale tutta la maggioranza, compreso il MoVimento 5 Stelle, al di là della questione della piattaforma, ha deciso come ha deciso. Vorrei però rivolgere un appello a tutti i colleghi, per ragionare ancora una volta su un punto.

Ho sentito parlare di primato della politica, del fatto che, in relazione a un programma elettorale, nel quale c'era scritto di bloccare i porti e di bloccare gli sbarchi, allora è giusto intervenire. No colleghi, attenzione, non è così, perché la democrazia è fatta di bilanciamenti: se si vogliono bloccare i porti

politica prevale su diritti costituzionali fondamentali come la libertà delle persone. Stiamo facendo questo ragionamento. Attenzione, c'è oggi e c'è domani, io non vorrei che questo precedente aprisse una questione. Voglio essere molto chiaro su questo punto: per me - l'ho sempre pensato anche in altre occasioni e lo ribadisco oggi con forza - il confronto e lo scontro politico sono sempre legittimi. Salvini è un dirigente politico, il Vice Presidente del Consiglio: per me va sconfitto politicamente e solo politicamente. Non ci può essere lo strumento della giustizia per una battaglia politica. Ma anche il contrario è valido: non ci può essere una ragione politica che prevale sulle leggi e sulla Costituzione. Questo è un problema molto serio, sul quale vi prego di riflettere. Noi non stiamo giudicando se il vicepremier è colpevole o no. Spetta ai tribunali, spetta al giudice la risposta a questo, non a noi. Sarebbe tuttavia assolutamente utile, per evitare che si aprisse un precedente pericoloso, che, coerentemente con le cose dette, si arrivasse a questo processo. Non voglio riprendere le affermazioni di principio fatte dai colleghi del MoVimento 5 Stelle nella loro storia di affermazione in questo Paese, ossia che tutti i cittadini sono uguali e hanno lo stesso diritto: non è questo quello che a me interessa in questo momento. Non vi pongo problemi di coerenza su ciò che è stato detto, su ciò che avete fatto, sui comportamenti che avete avuto rispetto ad altri che si sono trovati in vicende giudiziarie complesse. Io vi chiedo se ritenete davvero che, in nome di un'alleanza politica, si possa aprire quel precedente che riguarda tutti noi che non riguarda voi. Questa è la dimostrazione di una cosa che ho già avuto modo di sottolineare: «in nome del popolo» dice la Costituzione, ma il popolo attraverso le sue rappresentanze. Quando qualcuno parla in nome di tutto il popolo, di tutti i 60 milioni di italiani, per me, nell'esperienza della storia, è sempre un grandissimo problema, che attiene alla qualità della democrazia. Infine, consentitemi un'ultima considerazione. Il senatore Pillon ha detto: noi contrastiamo i mercenari, i delinquenti che speculano sulla vita delle persone.

Mi limiterò ad alcuni punti essenziali, pur sapendo bene che quello che dirò non cambierà la decisione della maggioranza, che ha il solo fine di mantenere in vita il Governo, non aiuterà a far cambiare idea nemmeno a coloro che hanno propagandato a lungo il cambiamento e, con esso, l'idea suggestiva che non ci sarebbe più stata alcuna immunità, né più privilegi per alcuno, senatori e onorevoli compresi. è infatti all'affermazione di un privilegio che si vuole approdare: un privilegio a cui, prima, il ministro Salvini ha dichiarato di volersi sottrarre, salvo poi ricredersi davanti alla necessità di conservare il potere, finendo così solo con il sottrarsi alla giustizia e al processo, attraverso il sostegno di un voto bugiardo della piattaforma Rousseau e, ancor peggio, dei più recenti richiami pubblici dei capi dei 5 Stelle - inaccettabili tanto nel tono quanto nel merito - con cui minaccia il deferimento ai probiviri per chi si azzarderà a votare contro l'oracolo o il responso della piattaforma della Casaleggio Associati. ai punti essenziali: in primo luogo la legge costituzionale ha qualificato come «insindacabile» la valutazione della Camera competente circa la sussistenza di una delle due famose esimenti. Tuttavia, la stessa Corte costituzionale ha specificato che l'insindacabilità può sussistere solo se la decisione assunta sia «congruamente motivata». Certamente la relazione che il presidente Gasparri ha presentato a nome della maggioranza è ampia e abbondante, quanto alla lunghezza delle considerazioni, ma solo a quella. A mio avviso, infatti, si rinvengono delle contraddizioni e, appunto, delle incongruità, che ne inficiano la sostanza argomentativa. Non voglio fare il causidico, la Consulta non ha parlato di conclusioni «adeguatamente motivate e lunghe», ma «congruamente motivate» e quindi plausibili, coerenti logicamente, giuridicamente non abnormi. Gli aggettivi contano in questo caso - eccome! - e su questo potrebbe giocarsi, in futuro, anche la partita di un eventuale conflitto di attribuzione. Non si tratta di un'insindacabilità illimitata: lo ha già detto la Corte più volte. nella relazione viene posta molta enfasi sulla tesi, forse un po' troppo creativa, circa il fatto che, in caso di irreversibili lesioni dei diritti fondamentali, nemmeno potrebbe essere ipotizzata la sussistenza di un reato ministeriale, potendosi trattare di un semplice reato ordinario. A dire il vero, tale principio non è mai stato affermato da nessuno in precedenza e non si può escludere, in linea generale ed astratta, che in particolari circostanze possa considerarsi ministeriale anche un reato che abbia prodotto tali conseguenze irreversibili. In ogni caso, condivisibile o no che sia questa tesi, però, allo stato, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che gli elementi che caratterizzano la categoria dei reati ministeriali sono «la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal Ministro, che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto» e non ha mai aggiunto altro. Lo Quindi, ravviso un primo sbandamento, che però rischia per la maggioranza stessa di essere un deragliamento vero e proprio. È evidente la strumentalità della tesi, che però va letta anche *a contrario*, nella sua terribile ammissione implicita. Intendo dire che nella relazione, in sostanza, si ammette che vi siano state lesioni di diritti fondamentali ancorché non irreversibili, altrimenti nemmeno si potrebbe ipotizzare il reato ministeriale. Ebbene, se la maggioranza ammette la lesione di diritti fondamentali, allora ne consegue - e non potrebbe essere diversamente - che il vaglio circa l'eventuale sussistenza di una delle due esimenti previste dalla legge deve essere particolarmente rigoroso, o, se si preferisce, che la preminenza dell'interesse pubblico perseguito deve essere particolarmente fondata e manifesta. Questo però non è avvenuto. Nella relazione, infatti, si esclude la sussistenza di un interesse personale - come sarebbe nel caso della ricezione di denaro per un atto d'ufficio ma anche di un interesse partitico, che, invece, rappresenta - non prendiamoci in giro - la vera finalità della condotta tenuta dal Ministro per essere al centro della scena politica e mediatica nella metà di agosto. La relazione è quasi apodittica e, comunque, carente nel motivare il preminente interesse pubblico perseguito. Il contrasto all'immigrazione clandestina? Affrontiamo allora il tema, che è estremamente complesso e non può essere ridotto a *slogan*. In questo senso, potrei far presente che non tutto il Paese è convinto che questo sia un preminente interesse pubblico. Vi sono state manifestazioni popolari di segno contrario e opinioni, anche di economisti, circa l'apporto degli extracomunitari non sarà un peccato se cito l'opinione del presidente dell'INPS Boeri sui contributi - per non voler citare i risultati non plebiscitari della piattaforma Rousseau e così via. Ma voglio scendere su quel terreno. Quella condotta è stata funzionale a tutelare quel presunto preminente interesse pubblico? Sappiamo benissimo che, alla fine, soprattutto delle persone trasferite nel Lazio si sono perse le tracce. Pertanto, quella condotta iniziale non è stata nemmeno concretamente funzionale a perseguire quell'interesse. Il cuore del problema è però forse un altro. La relazione ci gira intorno, ma tace su un punto decisivo. Non si dimostra, cioè, che «solo ed esclusivamente» con quella condotta - secondo la magistratura configura gli estremi del reato di sequestro di persona fosse possibile tutelare quel preminente interesse pubblico, non potendosi adottare alcun altro comportamento non configurante una fattispecie di reato. «Solo» mantenendo centinaia di persone in condizioni disumane e imbarazzanti sulla nave Diciotti, non facendole scendere e non indicando l'*hotspot* si è potuto tutelare l'interesse pubblico? E allora perché una condotta simile non era mai stata seguita dai precedenti Ministri? E allora perché l'uscente ministro Minniti, che pure ha conseguito indubbi risultati nel limitare l'arrivo di migranti nel nostro Paese, non ha avuto bisogno di ricorrere a questa modalità? Non si può arrivare all'assurda conclusione che solo con siffatte condotte possa esservi il contrasto all'immigrazione, con la conseguente conclusione che tutti i precedenti Governi, anche di centrodestra e pure con Ministri dell'interno della Lega, non avendole adottate, non hanno tutelato un preminente interesse pubblico.

e anche carenti, nella parte in cui non viene dimostrata l'esclusività funzionale della condotta contestata ai fini del perseguimento di quel supposto preminente interesse pubblico, che, tra l'altro, dovrebbe essere manifesto ed evidente e non oggetto di forti contrasti presso l'opinione pubblica. Ma, a ben guardare, nella relazione stessa si ha paura delle conclusioni affermate, laddove si specifica che non costituiranno un precedente vincolante, ma in futuro si dovrà sempre valutare caso per caso. E ci mancherebbe, dico io e direbbe anche *monsieur* Il problema sta nel metodo seguito, perché - questo sì - costituisce precedente, ovvero mascherare, a colpi di maggioranza, un interesse di partito di maggioranza, appunto - alla cui preminente tutela era in realtà rivolta la condotta contestata al Ministro dell'interno. Mi sia consentita

da parte dei dirigenti e, in particolare, del Ministero dell'interno. Sono state trasmesse lettere *ex post* del presidente Conte e dei ministri Di Maio e Toninelli, volte ad avallare la condivisione delle scelte operate dal fare attenzione perché la ministerialità del reato non era in discussione. La condivisione non sta a indicare, di per sé, la sussistenza di un preminente interesse pubblico. In termini tecnici, si tratta semmai di confessioni di aver concorso nel reato.

che il ministro Salvini sia per me già responsabile del reato di sequestro di persona: non lo so e nessuno di noi al momento può saperlo e quindi affermarlo. Restiamo garantisti, il che non significa però impunità, né sottrazione al processo. Intendo semplicemente ribadire che l'assenza di un'intuitiva evidenza nei termini indicati non può consentire l'attivazione di una guarentigia insopportabile, perché espressiva solo di una tutela politica dell'attuale

Voglio proprio guardarvi, colleghi, mentre lo fate. Voglio guardarvi tradire quel manifesto che, con presunzione, avete sempre affermato rendervi più onesti degli altri. Oggi dimostrate

Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, oggi ci troviamo in un ruolo un po' atipico: dobbiamo essere giudici di noi stessi. per quanto ci riguarda, la nostra bussola è la relazione del presidente Gasparri, al quale va il nostro plauso, perché puntuale e precisa, soprattutto per quanto concerne un punto, relativo alla tutela di interesse pubblico di rilevanza costituzionale di un organo costituzionale dello Stato, ossia il Governo della Repubblica. Vorrei partire dunque con delle domande retoriche,

Ha garantito loro la somministrazione di cibo e bevande? Sì. Ha garantito loro l'assistenza medica o sanitaria? Sì. E allora, che cosa c'è stato? C'è stata l'esigenza di trattenerli. Perché? Perché? Innanzitutto - e non solamente - perché andavano identificati, che penso sia una procedura necessaria per garantire la sicurezza del Paese: dobbiamo sapere chi entra in Italia e non è un dogma, è un'esigenza del popolo italiano. Vogliamo sapere chi entra nel nostro Paese, chi varca i nostri confini. C'è poi un tema di cui nessuno parla mai: è come quando si vuole prendere la polvere e la si vuole nascondere sotto il tappeto. Nessuno si preoccupa di dire dove andranno le persone una volta sbarcate. Ci si occupa solo di quando devono arrivare, di farle sbarcare e poi nessuno sa dove vanno, come campano e dove vivono e questo è un tema che non può essere ogni volta tralasciato, perché è fondamentale per la convivenza civile nel nostro Paese.

quindi, non vi è stata violazione di alcun diritto umano in quella circostanza. Vi è stata l'esigenza di condividere con altri Pesi europei un fenomeno di portata mondiale. E allora voglio dire con molta franchezza che ha fatto bene il presidente Gasparri quando ha ritenuto opportuno coinvolgere altri membri del Governo, perché l'atto

di questa compagine governativa. I problemi di siffatta natura non si risolvono a Lampedusa; non si risolvono nel Mediterraneo. Cari amici, questi problemi si risolvono a Bruxelles. Il problema è che, quando a Bruxelles si parla del fenomeno dell'emigrazione, un fenomeno storico mondiale, gli amici della Lega si astengono quando si tratta di modificare il Regolamento di Dublino e addirittura i 5 Stelle votano contro.

lottano per accedere ai servizi pubblici di non sentirsi discriminati. Questa è la vera sfida che abbiamo dinanzi a noi e non possiamo farlo con una visione manichea tra chi vuole e chi non vuole che entrino nel Paese gli immigrati.

Ieri abbiamo letto su un giornale che a Milano su 300 case popolari ben 215 sono state assegnate a degli extracomunitari. Queste vicende purtroppo generano

del Governo, colleghi senatori, colleghe senatrici, io non tratterò della vicenda sotto il profilo tecnico, perché già esaustivamente sono stati indicati, soprattutto nelle relazioni di minoranza, i limiti entro cui essa si svolge. È stato già detto che in questa sede dobbiamo limitarci a stabilire se all'epoca esistessero le condizioni per la tutela di quel particolare interesse dello Stato e, quindi, se tale interesse forse preminente rispetto ai diritti individuali che sono stati sacrificati nell'ambito della vicenda in esame, per sapere se esista e sussista l'esimente prevista dalla normativa vigente. Credo però che sia necessario mettere in luce il susseguirsi degli accadimenti, perché servono a chiarire quali siano le varie responsabilità. Intanto un dato che balza evidente agli occhi è che l'intera vicenda è impregnata di quelli che nelle aule giudiziarie vengono solitamente chiamati aggiustamenti processuali,

tra l'altro assunti in assoluta autonomia - come è stato confermato dalle persone sentite preventivamente e addirittura direi non solo in autonomia ma anche in solitudine - erano stati, secondo il contenuto di quelle lettere, concordati preventivamente dal Governo nella sua interezza.

Non è reperibile, infatti, in nessun luogo un atto del Governo dal quale risulti l'assunzione della decisione che ha originato l'intera vicenda, a meno che non dobbiamo credere che che essa sia stata assunta nel corso di qualche chiacchierata. Ma questo per gli atti di Governo è assolutamente impossibile. D'altro canto, giova anche rilevare che il presidente Conte, al di là di quanto anche ieri mattina ha dichiarato in quest'Aula, in quest'Aula, ha smentito se stesso, perché solo venti giorni prima aveva autorizzato lo sbarco - guarda caso - di immigrati dalla stessa nave Diciotti. Ripeto: solo venti giorni prima aveva, di autorità, ordinato lo sbarco, tra l'altro con il palese dissenso, reso pubblico, del ministro Salvini. Altrettanto deve dirsi per la lettera dei due ministri Di Maio e Toninelli, che corrono in soccorso per evitare che venga concessa l'autorizzazione e venga quindi messo in discussione l'intero impianto del Governo. Non esiste alcun atto formale del Governo e, tra l'altro, essi non solo smentiscono se stessi, ma svillaneggiano l'intero Movimento cui appartengono, che ha sempre sostenuto che le autorizzazioni a procedere vanno comunque Questo la dice lunga sulla coerenza e sulla genuinità della linea politica del MoVimento 5 Stelle, che adotta le proprie decisioni a seconda di chi siano i destinatari e secondo la convenienza del momento. Non basta: basta: è avvilente per quest'Assemblea aver letto e udito i messaggi che sono stati lanciati agli appartenenti al Gruppo, con cui sono state minacciate ritorsioni, nonché la segnalazione al collegio dei probiviri, ove non si attenessero alle indicazioni di voto della famosa piattaforma, che - com'è già stato detto ieri ieri - viene indirizzata dai grandi manovratori a seconda della convenienza. Un'altra tardiva linea difensiva, sfornita di fondamento, sfornita di fondamento, è data dal comportamento che avrebbero tenuto le autorità maltesi. Si è detto che in effetti la vicenda è nata perché le autorità maltesi avevano indirizzato la nave verso l'Italia, mentre in effetti era diretta verso Malta. Ebbene, a parte il fatto che questo attiene ad altro momento e ad altra vicenda, c'è da ricordare che, se ci

Si è detto anche che è stata assicurata l'assistenza sanitaria alle persone presenti e che erano stati riscontrati alcuni casi di scabbia. Ma anche questo è un clamoroso autogol che mortifica il diritto alla salute garantito dalla nostra Costituzione. Infatti, al di là del fatto che la nave era talmente piccola ed era impossibile assicurare assistenza adeguata a 177 persone, tra l'altro meritevoli di protezione da parte dello Stato, da parte dello Stato, se c'erano dei casi di scabbia credo che sarebbe stato doveroso far scendere immediatamente i malati, ricoverarli in ospedale e assicurarsi che avessero cure adeguate e soprattutto che il morbo non si diffondesse. Questo non è stato fatto.

Ma - vivaddio - se così era, non ci si può esimere dal complimentarsi con il Ministro dell'interno. Se fosse stato vero che esisteva un pericolo del genere, credo che un Ministro dell'interno adeguato avrebbe dovuto immediatamente, sull'imbarcazione stessa,

Questa è la condizione nella quale il nostro Ministro, con suo provvedimento, ha messo l'Italia.

Successivamente sono tornati indietro e hanno ritrattato questa versione.

mettendo a repentaglio la loro salute e anche la sicurezza nazionale, se è vero che c'era il sospetto che ci fossero tra loro dei terroristi. A questo punto è necessario concedere l'autorizzazione affinché il ministro Salvini si sottoponga al giudizio della magistratura che valuterà sull'esistenza o no delle responsabilità penali. Il Parlamento ne guadagnerebbe sicuramente in credibilità agli occhi del Paese, il sistema democratico ne trarrebbe giovamento e sicuramente ne uscirebbe anche rafforzato. Signor Presidente, è un tema delicatissimo quello che affrontiamo oggi per le implicazioni sul piano del diritto internazionale e del rispetto della nostra Costituzione. Sul piano del diritto internazionale mi limiterò alla sintesi assoluta fatta da Jürgen Habermas: una delle conseguenze del concetto di sovranità sviluppato dal diritto internazionale classico è il divieto di intromettersi in linea di principio negli affari interni di uno Stato internazionalmente riconosciuto. Nelle carte dell'ONU questo divieto viene confermato ma anche controbilanciato fin dall'inizio dallo sviluppo della tutela internazionale dei diritti dell'uomo. Prima conclusione: la sovranità non può mai, mai cancellare i diritti fondamentali dell'uomo. La legge costituzionale n. 1 del 1989 ha modificato l'articolo 96 della Costituzione proprio per superare i limiti precedentemente riscontrati ed ha adombrato uno stato di necessità politico-costituzionale capace di giustificare l'azione criminale di un Ministro. La riforma ha voluto sottrarre al Parlamento la qualificazione del fatto di reato e ha attribuito al Parlamento, in quanto organo politico rappresentativo, la funzione di poter inibire l'azione giudiziaria, a seguito del riscontro di interessi prioritari che emergono nel concreto dell'azione del Governo, i quali, in quanto permanentemente rilevanti per la collettività, potrebbero potrebbero venire soddisfatti anche attraverso il compimento di attività illecite. Ma questo è il nuovo articolo 96. Per questo, in dottrina, si dice che le Camere operano a difesa dei valori oggettivi della Costituzione. La normalità costituzionale: questo siamo chiamati a garantire. Vediamo di riassumere i fatti. Cominciamo con l'esercizio della sovranità. Ma quale Paese può ipotizzare di usare una propria nave militare, il suo equipaggio e 177 naufraghi salvati come ostaggi per una trattativa internazionale? Possiamo ritenerlo davvero un gesto proporzionato al fatto? Certo che no. Questa è una pagina che aggiunge solo discredito, se non anche disprezzo. La questione dirimente è, però, un'altra. Qual era lo stato di necessità che si era venuto a creare? Quale il pericolo per lo Stato? Gli interessi prioritari dello Stato permanentemente rilevanti, tali da consentire il compimento di attività illecite da parte di un Ministro? I 177 naufraghi? La nave Diciotti? Colleghe e colleghi, stiamo parlando della nave Diciotti e non del Bounty e dei suoi ammutinati. Una segnalazione di pericolo legato al terrorismo o alla sicurezza nazionale, all'ordine pubblico o a una possibile epidemia? Quale di questi elementi costituiva lo stato di necessità e il pericolo per lo Stato? Nessuno, perché al momento dello sbarco dei naufraghi e della liberazione dell'equipaggio della nave della Guardia costiera italiana nessun provvedimento amministrativo-giudiziario è stato emesso nei loro confronti. La realtà è che c'erano non fatti, ma solo atti politici; la volontà politica del Ministro di riaffermare la sua linea politica: i porti sono chiusi e non sbarca nessuno. Il principio essenziale del costituzionalismo consiste nella limitazione del Governo per opera del diritto. Questo ha voluto garantire la legge costituzionale n. 1 del 1989, riformando l'articolo 96, tendendo - come da dottrina prevalentissima - a rimarcare una funzione di carattere vigilatorio del Parlamento sull'operato politico dei Ministri, sottolineando così il ruolo del Parlamento quale supremo interprete dell'interesse pubblico e di quelli costituzionalmente rilevanti dello Stato. La convenienza politica del momento, l'ideologia politica del momento non possono calpestare la tutela della nostra Costituzione e cancellare i diritti fondamentali dell'uomo. Il principio democratico non è limitato al profilo della selezione democratica dei rappresentanti della sovranità popolare, ma ricomprende anche la garanzia dei valori fondamentali costituenti il contenuto dell'unità politica della Repubblica. Il Ministro dell'interno vuole mettere in discussione questa unità politica repubblicana, sposando la logica schmittiana della contrapposizione amico nemico. Sbaglia, soprattutto se, per farlo, pensa di poterlo fare infrangendo la legge. Sia la magistratura a decidere dell'operato del ministro Matteo Salvini e noi consentiamo che questo avvenga.

quello che noi siamo chiamati oggi a decidere può certamente segnare un momento, anche uno spartiacque nella nostra storia e, in qualche modo, nell'applicazione stessa della tante volte richiamata legge

a vedere la decisione assunta dalla Giunta, la strada sembra segnata - può costituire esattamente un precedente pericoloso, pericolosissimo e devo dire che la discussione e l'eco di alcuni interventi mi preoccupano ancor di più in tal senso. Ho sentito parlare

un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o un interesse pubblico preminente. Questa è la questione esatta su cui noi dovremmo pronunciarci. che bisogna mettere a confronto il bene tutelato dalla Costituzione e l'azione che è stata messa in campo, stabilendo se il fine era preminente rispetto al mezzo.

o di una linea cosiddetta di Governo? C'è un interesse di Governo che a questo punto si sostituisce, come già in qualche modo indicato dai relatori di minoranza come pericolo, a quello dello Stato costituzionalmente rilevante? Questo è il punto, ed è la questione che a me e a tutti noi preoccupa perché questo sì che diventerebbe un precedente pericoloso. Chiunque governa

non voglio usare parole forti, ma è evidente che lo scenario è quello - è se le azioni di Governo dei Ministri e del Presidente del Consiglio sono sciolte dalla legge, sono *legibus solutae*. È questo che stiamo affermando?

Certamente per me era fondamentale realizzare alcuni programmi, perché ognuno ha interesse a volerlo fare rapidamente per un interesse generale, come realizzare un grande parco, sistemare un'area protetta, far funzionare i

atti. L'ordine è stato dato verbalmente, c'è il mistero - non si capisce - di come e in quale forma sarebbero stati chiusi i porti;

di rispetto delle stesse leggi. Il punto è il seguente: il precedente che rischiamo con la decisione che stiamo per prendere in quest'Aula tra qualche ora è gravissimo.

quelle e sostituiscono l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, diventando di per sé interesse pubblico preminente. Ecco la questione grave che si rischia di affermare. È questo il precedente che a noi preoccupa

il PD e la sinistra vogliono processare il ministro Salvini per aver fatto il proprio dovere. Noi di Fratelli d'Italia pensiamo che dovrebbero essere processati molti dei suoi predecessori per non aver fatto il loro dovere. Coloro che oggi vorrebbero Salvini sul banco degli imputati sono gli stessi che, con la loro inerzia, la loro complicità, il loro ipocrita buonismo, hanno provocato l'invasione da parte di centinaia di migliaia di finti profughi. Un esercito di disperati, diventati in gran parte preda dello sfruttamento, del lavoro nero, della prostituzione, del traffico d'organi, e in altra parte, certo non meno rilevante, sono diventati manovalanza della criminalità organizzata, dello spaccio di droga e di ogni altro genere di traffico illecito. Solo chi si rifiuta di guardare in faccia la realtà può fingere di non vedere l'interesse pubblico nell'azione del Governo e del Ministro, volta a fermare il perverso intreccio tra scafisti e ONG, con queste ultime trasformate, consapevoli o no, in complici della tratta di esseri umani che, com'è noto, rende più del traffico di armi e di droga. C'è un dato che rende evidente l'interesse pubblico nell'azione del Ministro senza bisogno di tanti discorsi:

cento di furti. Quale sarebbe la colpa commessa dal Ministro nel combattere questa drammatica emergenza ereditata dai Governi del Partito Democratico? La colpa sarebbe - pensate un po' - avere impedito per qualche giorno lo sbarco sul suolo italiano dei naufraghi soccorsi dalla nave Come se la nave Diciotti non fosse un luogo sicuro, come se i naufraghi non fossero stati rifocillati e curati con tutte le attenzioni del caso.

«presi in carico e trasferiti in centri sorvegliati», come testualmente sancito del Consiglio europeo del 28 giugno, che tra l'altro ha raccomandato: «per «per smantellare il traffico di esseri umani ed evitare la tragica perdita di vittime umane è necessario eliminare ogni incentivo ad intraprendere viaggi pericolosi». È qui, cari qui, cari colleghi, che sta l'interesse pubblico. Chi arriva senza rispettare le regole, in Italia non deve essere considerato profugo fino a prova contraria: deve essere considerato clandestino fino a prova contraria. e quindi trattenuto fino al definitivo accertamento della sua reale condizione. E se non risulta avere diritto alla protezione (e questo lo dico anche al Ministro), deve essere espulso. Emigrare non è un diritto. Per fortuna, l'Italia non ha firmato il *global compact*, credo anche grazie all'opera svolta da Fratelli d'Italia in questo senso. se si dovesse muovere un rimprovero al Ministro sarebbe di non avere tenuto sotto controllo queste persone che sono sbarcate e averle lasciate scappare, come altre migliaia prima di loro. Ma questo non è il tema di oggi, che è invece l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. La sinistra ha ripetuto in quest'Aula, quasi come un ritornello, ritornello, che Salvini deve difendersi nel processo, non deve difendersi dal processo. Cari colleghi del PD che avete ripetuto questo ritornello tutta la giornata di ieri,

A noi e solo a noi compete accertare se sussista o no l'esimente speciale del preminente interesse pubblico. Non possiamo delegare questo compito alla magistratura, non è per legge sua competenza: o è una decisione che prendiamo noi, o è una decisione che nessun altro può prendere. Non si può dire di lasciare decidere il tribunale, occorre assumersi questa responsabilità e noi ce la assumiamo la responsabilità di affermare che l'interesse pubblico sussiste. Lo diciamo dopo aver studiato le carte e dopo aver letto la proposta del relatore, che condividiamo senza alcuna riserva. Lo diciamo senza nasconderci dietro un sondaggio come i colleghi del MoVimento 5 Stelle. Ma quale sondaggio? È come se il giudice, dopo aver ascoltato le conclusioni delle parti, nel dubbio se assolvere o condannare, sospendesse l'udienza e facesse una una consultazione con il pubblico, con il personale della cancelleria e con chi passa lì per caso. No, bisogna assumersi la responsabilità, noi siamo i giudici e noi di Fratelli d'Italia diciamo che non soltanto sussiste il preminente interesse pubblico, ma in questo caso sussiste un vero e proprio interesse nazionale, che è concetto e principio ancora superiore. Noi di Fratelli d'Italia, quando è in gioco l'interesse nazionale, sappiamo bene da che parte ci dobbiamo schierare.

UV))*. Signor Presidente, la scelta di oggi richiede da parte nostra un'assunzione di responsabilità fuori da ogni vincolo di partito, fuori da ogni ordine di scuderia. Tutti noi membri del Parlamento siamo chiamati a fare questa scelta in libertà di coscienza, ben sapendo che ogni nostra valutazione è, prima di tutto, di carattere istituzionale, riguarda l'equilibrio tra diversi poteri dello Stato e i margini di libertà che spettano alla decisione politica in uno Stato di diritto. Nei regimi illiberali tutto è controllato dal Governo, a partire dal potere giudiziario. Nei regimi antidemocratici - ne abbiamo un esempio nel Venezuela di oggi - non ci si può contrapporre al Governo. Nei regimi cosiddetti giudiziari, la sovranità della decisione dei magistrati non può essere discussa. Io rispetto, ovviamente, il parere di tutti, ha erroneamente ipotizzato che la valutazione che il Senato dovrà compiere oggi sul caso Diciotti debba essere incentrata su questa semplice domanda: può il mandato governativo conferito a un Ministro prevedere o no la commissione di reati? In realtà, tutti noi capiamo che, se questo fosse l'oggetto della nostra valutazione, sarebbe del tutto inutile e superfluo, in quanto in nessun caso un mandato governativo dato a un Ministro potrebbe prevedere *ex ante* la commissione di reati. La questione, invece, che siamo chiamati a valutare in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, articolo 9, comma 3 riguarda la circostanza se il Ministro abbia agito per il perseguimento di un interesse pubblico governativo o viceversa se abbia agito per una finalità inerente a un suo interesse privato. Questa, colleghi, non è la sede per esprimere valutazioni in ordine alla politica dell'immigrazione del ministro Salvini, perché questo giudizio noi lo abbiamo già espresso. Io personalmente l'ho espresso votando ripetutamente no ai voti di fiducia al Governo Conte. Nemmeno siamo chiamati ad esprimere un assenso o un dissenso sulla bontà dei provvedimenti adottati, ma solo sulla circostanza che queste decisioni siano state assunte per un interesse privato del ministro Salvini e non attuando scelte politiche concordate in sede di Governo e frutto di indirizzo politico. Dunque, colleghi, non sprechiamo l'occasione di una riflessione alta sullo Stato di diritto, in un'ulteriore tappa dell'infinita resa dei conti tra di noi. *(Richiami del Presidente).* Qui si tratta di difendere l'autonomia e la discrezionalità della politica e, così facendo, di difendere il principio che l'opposizione ai Governi è affidata al Parlamento e alle scelte dei cittadini, non al potere di supplenza accordato ai giudici. Mi consentano i colleghi del MoVimento 5 Stelle: oggi voi rinnegate una concezione in base a una cinica salvaguardia del Governo, non in base a una riflessione autocritica. Io faccio esattamente l'opposto: mi oppongo a questo Governo, ma non rinnego la mia concezione liberale, che affida agli elettori cittadini e non ai giudici il destino della nostra democrazia. Per questa ragione, voterò in conformità alla relazione Gasparri il no all'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'interno perché, in uno Stato di diritto, il suo destino viene affidato al voto degli italiani e non all'impropria supplenza esercitata dai giudici.

colleghi, altri in questi giorni e in questa lunga discussione hanno meglio di me illustrato le ragioni

un'emergenza e ponendosi l'obiettivo di governare il fenomeno delle migrazioni. Devo dire che, se questa è la linea del Governo, sul caso Diciotti e su molte altre vicende, non ultima quella di ieri, si è fatto il contrario. Non può essere certo definita un'emergenza la presenza di una nave di organizzazioni non governative con a bordo 177 persone, 177 disperati, tra cui donne e minori. Non può essere certo considerato un atto di governo dell'immigrazione pensare che si possa affrontare questo tema prendendo in ostaggio migranti salvati da organizzazioni non governative, lasciandoli in mare per poter condizionare l'Europa.

Ho l'impressione che lei, più che governare l'immaginazione, la stia usando per ragioni politiche. Lei ha montato, in questi mesi, un vero e proprio Truman *show*, in cui lei assegna le parti. Ci sono le ONG, che improvvisamente, da organizzazioni che aiutano a evitare le morti in mare, sono diventate i nemici da combattere;

il procuratore della Repubblica e, come ho visto stamattina, anche il magistrato giudicante, perché ha già deciso che bisogna mettere in carcere gli esponenti delle ONG, che ieri

150 persone e lei, nei dati del Ministero, ne richiama una sola e poi ne nasconde altre, ma ora ci arrivo. signor Ministro, vuole usare il tema politicamente, per fare propaganda e per presentarsi come l'uomo dei porti chiusi, capace di illudere gli italiani che sta cancellando un fenomeno epocale, come quello dell'immigrazione. Lo sta facendo mostrando la faccia feroce e la faccia cattiva, trattando male un po' di disperati per disincentivare gli sbarchi di persone, che attraversano deserti e si mettono in mare rischiando la vita. Se però mostriamo la faccia cattiva - così mi è stato spiegato, quando abbiamo discusso il decreto sicurezza - non partono più. Questo però non sta succedendo

Se vuole fare l'interesse preminente del Paese, deve affrontare la realtà. È vero: non c'è alcuna emergenza dalla Libia.

che in un anno sono sbarcate, con piccole barchette a vela, governate da organizzazioni italiane e straniere, 7.000 persone, con 200 sbarchi, e questi sono solo i dati arrivati sul tavolo delle Procure.

Entrano di nascosto, gestiti da organizzazioni anche italiane, che li portano a destinazione. Quando il Ministro dell'interno comincerà a spiegare che questo è il problema? Quando il Ministro dell'interno, invece di prendersela con i poveracci della Diciotti o della barca di ieri o con le ONG, comincerà ad elevare un allarme e metterà in campo interventi? Parliamo

So che dire queste cose, signor Ministro, rischia di distruggere la sua immagine di uomo forte e coraggioso, che ha blindato le frontiere. È facile accanirsi su qualche disperato, ma è più difficile mettere in sicurezza il Paese, che ha 4.000 chilometri di coste, in cui si sbarca a Marsala, a Lampedusa o a Trapani.

perché io conosco un popolo che con lei non è d'accordo. Noi pensiamo che non possano essere le 200.000 persone che hanno manifestato a Milano a decidere se le sue azioni sono state legali o illegali,

Signor Presidente, illustri membri del Governo, colleghi senatori, partirò dai fatti, sapendo che in politica, come nella vita, i fatti si prestano a interpretazioni, vanno calati in un contesto e spesso danno origine a conseguenze che nulla hanno a che vedere con la loro natura. Politicamente parlando, i fatti che riguardano la vicenda della nave Diciotti rappresentano un disastro politico da ogni punto di vista. È disastrosa l'immagine di un Governo che vieta a una nave della Marina militare di attraccare in un porto nazionale disastrose sono le conseguenze politiche. Tre furono le premesse fatte dal Ministro dell'interno: l'Europa dovrà farsi carico dell'accoglienza dei migranti trasportati dalla nave Diciotti; la nave non attraccherà in un porto italiano; nessun migrante toccherà il suolo italiano. L'Europa, come d'abitudine, non si è fatta carico dei migranti della nave Diciotti, così come non si è fatta mai carico dei migranti che attraversano il Mediterraneo per accedere in Europa attraverso la porta più vicina, più vicina, che - disgraziatamente - è quella italiana. La nave «Diciotti» ha attraccato in un porto siciliano e tutti i migranti sono scesi su suolo italiano. La vicenda è stata resa quanto mai urticante anche in ragione del fatto che lo stesso Viminale ha spiegato che il divieto di attracco per la Diciotti era giustificato con il sospetto che su quella nave potessero essere stati imbarcati dei terroristi. Se erano terroristi, li abbiamo liberati sul nostro territorio nazionale. Questi sono i fatti, i fatti, che però sono stati interpretati, legittimamente, in maniera opposta alla loro natura, perché si collocano in un contesto in cui lo Stato - non la persona fisica Matteo Salvini, ma la funzione che Matteo Salvini ricopre cerca, come meglio può, di contrastare la pretesa di organizzazioni non governative di aprire di fatto un corridoio umanitario, spesso trasportando direttamente dalle coste libiche verso le coste italiane migliaia di migranti. Ciò avviene a fronte di un fenomeno che, con tutta evidenza, è epocale e incide su un Occidente che, proprio in questa fase storica, ha smarrito la propria identità a causa della globalizzazione, del cambiamento del contesto e del sistema di vita e di tanti altri fenomeni, non ultimo la sistematica desovranizzazione degli Stati nazionali, che è poi all'origine dei fenomeni politici cui stiamo assistendo non solo in Italia, ma in tutta Europa. Mi rendo conto del fatto che la parola «identità» non dica molto alla sinistra, che è cresciuta con il mito, evidentemente fallito, del multiculturalismo. Mi rendo conto che dica poco anche alla sinistra rappresentata dal MoVimento 5 Stelle, che ha in Jean-Jacques Rousseau il proprio nume tutelare.

la Chiesa e la religione che si possono permettere il lusso dell'etica dei princìpi, cioè a dire si fa quel che si ritiene giusto indipendentemente dalle conseguenze che le azioni presuppongono. Ma persino un uomo di chiesa come Papa Francesco ha legato l'accoglienza dei migranti alla possibilità concreta di integrare i migranti nella società italiana, possibilità che con tutta evidenza lo Stato italiano non riesce ad assolvere, ammesso che siano poi tutti integrabili in egual misura. Un paio di anni fa ho commissionato un sondaggio ad un autorevole sondaggista, Antonio Noto, poi pubblicato su «Quotidiano nazionale», per cercare di capire come effettivamente i musulmani residenti in Italia, quelli che si ritiene siano già integrati, ragionino, vivano e pensino il loro essere in Italia. Ebbene, i dati sono stati piuttosto sconcertanti. Il 31 per cento dei musulmani residenti in Italia ritiene che le donne non abbiano gli stessi diritti degli uomini e debbano portare il velo; il 41 per che le donne non debbano studiare e non debbano emanciparsi attraverso lo studio; il 25 per cento ritiene che le donne non debbano neanche guidare l'automobile. Il 58 per cento si dichiara non integrato - e questo evidentemente è un fallimento dello Stato per cento del totale dichiara di non volersi integrare e questo per lo Stato è un problema, un problema che ritengo che uno Stato e chi *pro tempore* ne rappresenta le funzioni ha il dovere di contenere. Pertanto l'azione del Governo rispetto alla vicenda Diciotti, calata in questo contesto, è un'azione legittima, che legittimamente interpreta un interesse pubblico e questo non credo sia contestabile. Se oggi ne stiamo parlando con questa gravità, se si è sfiorata una crisi di Governo su questo è perché veniamo da venticinque anni di sistematica delegittimazione della politica e della funzione politica, nonché della differenza che il politico rappresenta rispetto al comune cittadino. Abbiamo modificato articoli della Costituzione che prevedevano quello che oggi è di moda definire il primato della politica: dall'abolizione dell'immunità parlamentare all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, alla legge Severino, fino alla discutibilissima legge sul traffico di influenze illecite, non abbiamo fatto altro che delegittimare in radice la politica, impedendo così alla politica di manifestarsi per quello che effettivamente è. Da qui il trauma che stanno vivendo i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che sono cresciuti con quella retorica, su quei presupposti, attorno a quei princìpi che nulla hanno a che vedere con l'etica delle responsabilità, tant'è che sistematicamente li stanno mettendo in discussone, contravvenendo alla loro identità, ma così passando dall'età adolescenziale all'età adulta. Credo che sia dunque un processo utile nel quadro della maturazione della democrazia rappresentativa. Sorprende che a mettere in discussione questo principio sia stato lo stesso Matteo Salvini nel momento in cui, all'inizio della vicenda Diciotti, ha detto che si sarebbe fatto giudicare. E allora, se persino al ministro Salvini sfugge la differenza tra l'uomo e la funzione che l'uomo ricopre, tra il *leader* politico e lo Stato con le sue prerogative, a maggior ragione ritengo che ci sia il dovere da parte nostra e di quest'Assemblea di affermare il principio e quindi di difendere, non la persona fisica Matteo Salvini, ma le funzioni che quella persona ricopre, oserei dire indipendentemente e nonostante chi in quel momento la rappresenta. Grazie.

l'Assemblea è oggi chiamata a pronunciarsi in merito alle conclusioni della Giunta, in relazione alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini formulata dal tribunale dei Ministri. *In primis*, vorrei soffermarmi sugli sviluppi dei lavori della Giunta. I componenti di quest'ultima hanno deliberato a maggioranza l'approvazione della proposta del Presidente, recante nel dispositivo il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. La ragione di tale decisione prende le mosse da quanto disposto dalla legge di attuazione dell'articolo 96 della Costituzione, la legge costituzionale n. 1 del 1989, che, all'articolo 9, comma 3, prevede che, nell'ambito dei procedimenti aperti nei confronti dei Ministri, l'Assemblea possa, a maggioranza assoluta dei componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero al fine di perseguire un preminente interesse pubblico. In via preliminare sarebbe necessario quindi effettuare un parallelismo tra le richieste di autorizzazione a procedere formulate in relazione all'articolo 68 e quelle che discendono dall'articolo 96, così come interpretato dalla legge costituzionale n. 1. L'autorizzazione al procedimento penale contro i Ministri non verte intorno al cosiddetto *fumus persecutionis*, che, viceversa, costituisce l'oggetto della valutazione rimessa alla Camera competente *ex* articolo 68 Ciò in linea con l'intento di riporre integralmente nelle mani dell'autorità giudiziaria ordinaria le valutazioni di carattere strettamente giuridico concernenti la *notitia criminis*, rimesse interamente al Tribunale dei ministri. Di converso, la verifica delle finalità rappresentate dalle scriminanti previste dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. l del 1989, costituiscono l'oggetto di una scelta politica sottratta alla libera valutazione del giudice. Un profilo ulteriore di evidente distanza tra i due dettati si sostanzia nella forma attraverso la quale si arriva all'eventuale pronuncia del diniego. Infatti, a differenza di quanto previsto dall'articolo 68 della Costituzione, vale a dire un procedimento a forma libera, l'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 vincola il pronunciamento del diniego all'autorizzazione al riscontro di parametri espressamente individuati: l'aver agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Se ne deduce che la Camera di appartenenza debba considerare un dovere imprescindibile votare a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere nei casi in cui non vengano riconosciute alternativamente le scriminanti ivi previste ad un reato ministeriale. *A contrario* si potrebbe affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che nei casi in cui l'Assemblea ravveda nelle condotte poste in essere da un Ministro gli estremi di concessione di una delle scriminanti sopra esposte, questa sia obbligata a negare l'autorizzazione a procedere anche in quei casi in cui l'azione del Ministro possa aver sacrificato altri beni ordinariamente protetti dalle norme penali. Ovviamente il tutto con le dovute limitazioni. Infatti, l'autonomia della funzione di Governo, in relazione alle condotte che hanno ingenerato il procedimento a carico della parte, dovrebbe muoversi nell'ambito della valutazione della precondizione inerente alla ministerialità del reato. In questa fase si collocano, sul piano sistematico e procedurale, le riflessioni circa la non configurabilità dei reati ministeriali in relazione a fattispecie criminose che ledano in modo irreversibile determinati diritti fondamentali. Infatti, un omicidio di Stato non sarebbe mai configurabile nel nostro ordinamento costituzionale, non superando il vaglio preliminare circa la ministerialità del reato e venendo quindi a ricadere nell'area dei cosiddetti reati comuni, sottratti in quanto tali sia alla competenza del tribunale dei Ministri sia al filtro dell'autorizzazione a procedere della Camera competente. Ai fini della configurabilità della scriminante prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 occorrerebbe, invero, rendere edotta codesta Assemblea di come anche autorevole dottrina interpreti le due scriminanti ivi previste. Orbene, mentre la prima (l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante) fa riferimento a interessi che la stessa Costituzione considera come fondamentali per la vita dello Stato, la seconda (il preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo) si differenzia dalla prima perché legata non più all'interesse, bensì alla funzione. Nel caso che ci compete ci troviamo proprio dinanzi a quest'ultima prospettiva ed in questa ipotesi la riduzione dell'arbitrio insito nell'ammettere il sacrificio di beni protetti dalla norma penale, dinanzi all'esigenza di tutela dell'azione di Governo, richiede che l'area del politicamente preminente venga circoscritta, dal richiamo al costituzionalmente rilevante, sia pur indirettamente ed in modo meno evidente rispetto alla prima delle due ipotesi giustificative ora in esame. Il nostro ordinamento ammette delle cautele affinché vi sia una opportuna valutazione dell'attività di Governo in relazione alla tutela dei valori essenziali per l'interesse generale. accorgimenti fanno sì che la scriminante in esame non possa essere volta al conseguimento di meri interessi politici di parte, ovvero alla salvaguardia di un interesse personale del soggetto che se ne avvale. cautele sono la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, richiesta per avvalorare la decisione di esprimere il diniego all'autorizzazione, l'obbligo di motivazione della relazione della Giunta. Fatta questa necessaria premessa, è il caso di esporre la fattispecie che ci compete. Il ministro Salvini è stato ad oggetto di una richiesta di autorizzazione a procedere per il delitto di sequestro di persona aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, dall'abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per aver commesso il fatto anche in danno di soggetti minori di età, con riguardo alla nota vicenda giudiziaria circa la permanenza a bordo della nave della Guardia costiera Diciotti di 177 migranti. Occorrono diverse precisazioni. La prima verte su una corretta qualificazione dell'azione del Ministro in relazione al preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. La seconda muove da un corretto bilanciamento tra la condotta posta in essere dal Ministro e gli interessi lesi dalla stessa. Mettendo in evidenza l'agenda politica del periodo di riferimento, si evince in maniera chiara che l'azione del Ministro sia stata volta alla salvaguardia del preminente interesse pubblico in relazione all'azione di Governo. E questo in rapporto ai diversi impegni istituzionali, sia in ambito nazionale che europeo, al fine di rendere necessaria una comune assunzione di responsabilità del problema della gestione dei flussi migratori, sollecitando una più equa redistribuzione dei migranti in ambito europeo. Si può citare infatti quanto affermato dal Presidente del Consiglio, il quale in data 5 giugno 2018, in sede di dichiarazioni programmatiche, dinanzi all'Assemblea del Senato ha auspicato il superamento del Regolamento di Dublino al fine di ottenere l'effettivo rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità, di realizzazione di sistemi automatici di ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo, di riorganizzazione del sistema di accoglienza e di sottoscrizione di accordi bilaterali con Paesi terzi per la gestione dei flussi migratori. In sede di comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno del 2018, il presidente Conte, nel corso della seduta del Senato svoltasi il 27 giugno, ha individuato una serie di obiettivi volti: ad un superamento del criterio di primo arrivo, per mezzo dell'affermazione del principio secondo il quale chi sbarca in Italia sbarca in Europa; ad un'assunzione di responsabilità comune europea nei confronti dei salvataggi in mare; alla creazione dei centri di accoglienza in più Paesi europei volti a un corretto bilanciamento tra i diritti di chi arriva, da una parte, e la salvaguardia dell'ordine pubblico dall'altra. Le comunicazioni del presidente Conte, in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, hanno avuto ad oggetto la gestione condivisa multilivello dei flussi migratori, in modo tale da privilegiare un approccio strutturale rispetto ad uno emergenziale, chiedendo una risposta comune già nelle fasi di sbarco e, in seguito, di redistribuzione e rimpatrio senza oneri aggiuntivi per i Paesi di primo arrivo come l'Italia. Infine, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018, svoltesi al Senato l'11 dicembre, il Presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di dare corpo a una regolazione e gestione dei flussi migratori di matrice autenticamente europea. Inoltre, l'indirizzo governativo sulla vicenda Diciotti è stato espresso nella seduta dell'Assemblea del 12 settembre 2018. In ultimo, è utile ricordare che nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione a procedere in Giunta sono stati acquisiti, come allegati presentati dal Ministro dell'interno, atti che portano la firma del Presidente del Consiglio, del Vice Presidente Di Maio e del Ministro delle infrastrutture che muovono nella stessa direzione rispetto a quella prospettata dal ministro Salvini. Chiarito che il perseguimento di un interesse pubblico governativo ha caratterizzato nelle sue finalità il comportamento del ministro Salvini, occorre procedere ad escludere che il diritto leso sia un diritto incomprimibile e, in subordine, a un corretto bilanciamento tra la condotta posta in essere, da una parte, ed i beni giuridici lesi dall'altra. È indubbio che i migranti in questione siano dovuti rimanere a bordo della nave Diciotti cinque giorni in più a causa della mancata autorizzazione allo sbarco. Tuttavia, tale nave poteva considerarsi luogo sicuro, essendo ancorata in porto ed essendo costantemente assistita da medici e rifornita di generi di prima necessità. menzionato il fatto che i naufraghi in precarie condizioni fisiche e i minori non accompagnati erano già stati fatti sbarcare. Va altresì evidenziato che, una volta discesi a terra, i migranti in questione non sarebbero stati liberi di circolare sul territorio italiano, ma sarebbero stati accompagnati nei centri *hot spot*, a norma del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, per le procedure di identificazione. In altre parole, il diritto compresso nel caso di specie non sembra essere quello della libertà personale *tout court*, bensì piuttosto quello della libera circolazione. In ogni caso il diritto degli stranieri ad accedere e circolare sul suolo italiano non è un diritto assoluto ed inviolabile potendo prevedere compressione a fronte del diritto-dovere dello Stato di identificare gli stranieri e disciplinarne e limitarne gli accessi. Lo stesso articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, infatti, prevede la possibilità della compressione del diritto fondamentale della libertà personale per impedire gli accessi illegali nel territorio di uno Stato straniero. Se è vero che tale articolo prevede che dette detenzioni debbano essere regolari ed ove si ritenga che la "detenzione", verificatasi nel caso di specie, sarebbe avvenuta al di fuori di una disciplina legale prestabilita, cionondimeno la mancanza di norme che consentano il ritardo dello sbarco rileva al solo fine della verifica dell'eventuale illegalità della condotta del Ministro, ma non anche dell'indagine circa la natura del diritto compresso che il predetto articolo 5 non considera evidentemente come assoluto, prevedendone fisiologici casi di limitazione. Escluso dunque che i diritti compressi nel caso di specie possano annoverarsi tra i diritti fondamentali per così dire "incomprimibili", occorre infine effettuare il bilanciamento tra l'interesse perseguito e il sacrificio imposto ai predetti diritti dei singoli. A tal fine, occorre rilevare come il tempo trascorso a bordo della nave non si sia protratto oltre il tempo strettamente necessario al Governo per affrontare la questione del ricollocamento dei migranti in Europa e in altri Paesi extra Unione europea. Non sono noti specifici danni subiti dai naufraghi a causa di tale attesa, considerata anche la costante assistenza loro riservata a bordo e l'intervenuta autorizzazione allo sbarco per minori non accompagnati e soggetti in precarie condizioni fisiche. Il rinvio dello sbarco è stato peraltro correlato all'attesa del vertice europeo fissato per il 24 agosto, sicché è risultato proporzionato rispetto all'iniziativa comunitaria intrapresa. Con ciò non si vuol disconoscere l'eventuale disagio provocato ai migranti trattenuti a bordo della nave, molti dei quali sicuramente già provati da precedenti sofferenze, nonché dalla tragedia stessa della migrazione. Si ritiene tuttavia che vi sia stato, nel caso di specie, un adeguato bilanciamento tra tale disagio e gli importanti obiettivi perseguiti dal Governo. Prova ne sia che l'autorizzazione allo sbarco fu comunque concessa il 25 agosto senza ulteriori attese, nonostante l'esito non favorevole dell'incontro europeo Vista l'insussistenza della compressione di diritti assoluti e l'assenza di accertati danni fisici e psichici conseguenti all'azione del Ministro, si ritiene dunque che gli interessi pubblici perseguiti nel caso di specie possano ritenersi preminenti rispetto al sacrificio costituito dal trattenimento a bordo di una nave, in cui i migranti non sono stati coartati a salire, ma in cui anzi hanno trovato salvezza rispetto al proprio naufragio, per un tempo limitato

non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona ma lo faccio assolutamente tranquillo e sereno. Amo il mio Paese e da nove mesi dedico ogni mia energia a difendere la sicurezza, i confini e la serenità degli italiani, quindi ritengo un mio privilegio raccontarvi cosa è successo. Con l'intervento in quest'Aula intendo sottoporvi alcuni elementi di valutazione che reputo essenziali per chiarire ogni aspetto della vicenda Diciotti, visto che ho ascoltato parecchie inesattezze. La procura La procura della Repubblica di Catania, in conformità con quanto disposto dal tribunale dei ministri, ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei miei confronti, trasmettendo gli atti relativi. Sottolineo innanzitutto che non sono stato io a sollecitare la trasmissione degli atti. Qualcuno forse non ha capito che per andare a processo dovrei mentire a questo Senato e agli italiani e dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico del mio Paese e a me dire le bugie viene poco e viene male, soprattutto in un'Aula come questa. È un mio limite, perdonatemelo. atti. Venuto a conoscenza della esistenza d'indagini, ho atteso le valutazioni del tribunale restando a disposizione dell'autorità giudiziaria e astenendomi anche dal depositare atti e memorie volti ad ottenere il riconoscimento della natura ministeriale del reato che mi si contesta. Cinque diversi uffici giudiziari hanno autonomamente ravvisato la natura ministeriale delle condotte attribuitemi, e di tale circostanza non posso che prendere atto. Spetta ora al Senato valutare se il Ministro dell'interno abbia agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante dello Stato ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione oggi. Mi limiterò, per parte mia, a ricostruire in modo corretto ed esaustivo quanto avvenuto, perché è essenziale chiarire che la vicenda Diciotti non inizia con l'attracco della nave al porto di Catania, ma molto prima. Dalla ricostruzione dei fatti delle Forze dell'ordine, emerge che si è in presenza di un'iniziativa del Governo italiano coerente con la politica relativa ai flussi migratori. Perdonatemi, io di solito non mi emoziono quando parlo, ma c'è di mezzo

io abbia fatto privatamente, abusando della mia carica, qualcosa che ho fatto, faccio e farò per difendere la sicurezza dei miei e dei vostri figli, perdonatemi un po' di emozione. *(Applausi dai I numeri dicono che, così facendo, abbiamo salvato migliaia di vite: 2015: immigrati sbarcati 153.000, vittime recuperate in mare 296; 2016: immigrati sbarcati in mare 181.000, vittime recuperate in mare 390; 2017: immigrati sbarcati 119.000, vittime recuperate in mare 210; 2018: immigrati sbarcati 23.370, vittime recuperate in mare 23; 2019, a ieri: immigrati sbarcati 348, vittime recuperati in mare una. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti. Questi sono i dati. Più che dei porti aperti, qualcuno era sostenitore dei cimiteri aperti e non è la mia fattispecie: meno partenze, meno sbarchi, meno morti. Come anticipavo, è essenziale la genesi della vicenda. Il centro coordinamento soccorso marittimo della Capitaneria di porto italiana veniva informato, il 14 agosto scorso, dell'avvistamento in acque libiche di un natante con numerose persone a bordo che faceva rotta verso Malta: Il 15 agosto il natante si trovava nella zona di competenza del centro coordinamento soccorsi di Malta, che assumeva il coordinamento dell'evento. Alle 10,35 Malta comunicava all'Italia che, al momento, si stava limitando a monitorare lo stato del natante. Successivamente, due imbarcazioni maltesi inducevano il natante a deviare la rotta in direzione Italia. Tali circostanze oggettive sono confermate, in atto, dalle dichiarazioni rilasciate, peraltro, anche da uno dei presenti sul barcone, che dichiara: i maltesi hanno espressamente detto che non ci avrebbero mai condotto a Malta. Ci hanno seguito e ci hanno abbandonato in direzione Italia, facendoci cambiare rotta. Ditemi voi se è un comportamento degno di un Paese membro dell'Unione europea, che poi fa le lezioni a qualcun altro. Di Europa, però, riparleremo il 26 maggio. Sul punto, può essere chiarificatrice la testuale ricostruzione dei fatti del tribunale dei Ministri di Palermo. Il dirottamento (si parla addirittura di dirottamento) imposto dai maltesi, all'evidente fine di spingere il barcone in acque italiane, ha comportato un considerevole allungamento della traversata in quanto, invece di cinquanta miglia, ne hanno dovute percorrere percorrere cento. E la nave Mare Jonio, che ha fatto esattamente la stessa cosa tra Libia e Italia (mettendo a rischio la vita delle persone che pensano di aver salvato), è esattamente una fattispecie simile.

perché noi soccorriamo tutti e perché io non sarò mai il Ministro, l'uomo o il membro del Governo che lascia morire senza muovere un dito una sola persona del mar Mediterraneo: mai una sola persona. Questo sia chiaro a tutti. Abbiamo salvato. Abbiamo soccorso. Abbiamo curato. Abbiamo nutrito. Abbiamo aperto un contenzioso: acque di un altro Paese sovrano, impegni assunti in sede di Consiglio europeo.

la notizia del processo, l'Irlanda, l'Albania, la Conferenza episcopale italiana e altri Paesi europei. È chiaro ed evidente, infatti (ed è agli atti) che quei quattro giorni di permanenza in un porto italiano in attesa di sbarco, avendo fatto scendere tutti quelli che dovevano scendere, sono serviti, nell'interesse pubblico italiano e rispettando i dettami della Costituzione che parla di una sovranità del nostro Paese in caso di inadempienze da parte degli altri, a svegliare qualcuno che, evidentemente, stava dormendo. Quindi, quei quattro giorni sono stati risolutivi, ma non abbastanza per qualcuno, evidentemente. Aderendo a una richiesta del 19 agosto (e c'è una nota verbale, non sono parole: è tutto per iscritto), il Direttore generale affari interni della Commissione europea ha convocato, per il 21 agosto successivo, una riunione (tenutasi tre giorni dopo, il 24 agosto) e in quelle ore si è risolto il problema, senza esporre ad alcun rischio gli ospiti della nave Diciotti. Volevamo coinvolgere la comunità internazionale che, fino a un mese prima, non muoveva un dito e ci siamo riusciti. E i numeri che vi ho portato a testimonianza prima mi sembra siano evidenti. Addirittura, la Capitaneria di porto, per iscritto, aveva parlato di una guerra con Malta. Quindi, più interesse pubblico nazionale, più rispetto dei diritti previsti dalla Costituzione italiana in questa fattispecie non si potevano esercitare, dal mio punto di vista. Ribadisco il fatto che la Diciotti ha attraccato a Catania; questo fatto non può sovvertire il principio giuridico della responsabilità e degli oneri di primaria accoglienza in capo ad altri, come abbiamo sempre fatto noi. Solo all'esito della riunione, alla fine convocata, la Capitaneria di porto ha avanzato formale richiesta di porto sicuro, sollecitamente rilasciato, e, nella notte tra il 25 e il 26, i migranti sono stati sbarcati per poi essere trasferiti via terra all'*hotspot* di Messina. Nelle more della conclusione della trattativa, lo Stato italiano ha inoltre avviato contatti ad ampio raggio per coinvolgere altri Paesi nella redistribuzione degli immigrati, come previsto non sono nel contratto di Governo, ma anche nel programma di Governo e nel buon senso che è insito in ciascuno di noi. L'intera ricostruzione è del tutto in linea con le osservazioni del procuratore della repubblica di Catania, che tengo a ringraziare perché proprio oggi, mentre noi siamo qua a discutere, grazie all'azione congiunta di Forze dell'ordine e magistratura, sono stati compiuti 14 arresti di membri di un *clan* mafioso per traffico di droga

Lo stesso procuratore della Repubblica di Catania sottolineò come nella vicenda che mi riguardava sia stato esercitato un potere nell'interesse pubblico nazionale, come tale insindacabile da parte di un giudice penale. Questo è agli atti. Va poi osservato che gestione, monitoraggio e controlli dei flussi migratori appaiono ovviamente strettamente connessi all'interesse nazionale, sussistendo anche chiari profili attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla sicurezza della Repubblica, come del resto sottolineato dal direttore generale del Dipartimento informazioni per la sicurezza, che il 13 giugno 2018 sottolineò la centralità assoluta della minaccia jihadista nell'agenda di sicurezza di tutto il mondo. In questo contesto non deve neppure essere sottovalutata la possibilità che i flussi migratori possano rappresentare il veicolo per l'arrivo in Italia di soggetti infiltrati allo scopo di compiere azioni violente. Cito a titolo esemplificativo solo tre casi di specie che riguardano il cittadino bengalese Yasin Khan, sbarcato in Italia nell'ottobre 2016 dalla Libia, successivamente collocato in una struttura di accoglienza del bresciano, poi indagato per apologia del terrorismo e sottoposto a custodia cautelare in carcere; sottolineo il caso del cittadino gambiano Landin Touray, sbarcato nel nostro Paese nel 2017, residente in una struttura di accoglienza per richiedenti asilo nei pressi di Napoli, che ha prestato giuramento di fedeltà al Califfato, sospettato di appartenenza allo Stato islamico; da ultimo ricordo il caso del cittadino gambiano Sillah Osman, sbarcato dal Mediterraneo, richiedente protezione internazionale e e arrestato per il reato di partecipazione all'organizzazione terroristica denominata Stato islamico. È chiaro quindi che la questione dei flussi migratori e la gestione dei flussi migratori, in particolar modo quelli provenienti dalla Libia e dalla Tunisia, rivestono evidente attinenza con la sicurezza, l'ordine pubblico e la tutela dell'ordine pubblico nel nostro Paese, che sono competenze di spettanza di un Ministro dell'interno, non geniale, ma normale. Desidero confermare a quest'Aula, in conclusione, che il Governo di cui mi onoro di essere vice presidente e ministro dell'interno ha sviluppato fin dal suo insediamento con chiara e unanime determinazione

Collina)* - misure e azioni volte al contrasto dei flussi migratori irregolari e del *business* del traffico degli esseri umani del Mediterraneo che, secondo i servizi di *intelligence*, era arrivato a rendere più del traffico di droga e del traffico di armi. Quindi chi sta collaborando allo stroncare il traffico di esseri umani sta dando una mano anche a coloro che combattono il traffico di droga e di armi, perché il *business* dell'immigrazione clandestina proprio in armi e droga reinveste i suoi proventi e io e il Governo di cui mi onoro di far parte non saremo mai complici dei trafficanti di droga e dei trafficanti di armi. Questo sia chiaro ed evidente a tutti. I risultati dell'azione politica decisa di questo Governo sono sotto gli occhi di tutti: basta saper leggere i numeri. Si tratta di una dinamica straordinariamente positiva, sintomatica di un'inversione strutturale di tendenza, favorita da scelte adottate sia sul versante interno che sul versante internazionale. L'esecuzione del salvataggio da parte dell'Italia, come detto, in zona SAR maltese avrebbe comunque dovuto obbligare quello Stato - come in altre occasioni - ad assumere la responsabilità dell'evento e ad accogliere gli immigrati. Osservo che lo Stato italiano, pur intervenendo in via sostitutiva per salvare gli immigrati da un naufragio certo e garantire loro ogni pieno livello di assistenza, ha portato finalmente all'attenzione dei *partner* europei le problematiche connesse alle operazioni di di salvataggio e recupero e ai loro seguiti. Ciò nell'ambito di una controversia internazionale che doveva essere portata a immediata soluzione, nel legittimo esercizio della propria sovranità nazionale

soluzione nel legittimo esercizio della propria sovranità e nel quadro della parità e del pieno rispetto dei princìpi di solidarietà insiti nei rapporti di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea. Non posso, infine, sottacere che l'azione attuativa dell'indirizzo governativo in materia, sottolineata dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte nell'informativa del 12 settembre scorso a questa Assemblea del Senato, costituisce di per sé l'evidenza di un preminente interesse pubblico, rappresentato dalla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, che sarebbero stati messi a repentaglio - e saranno messi a repentaglio - in caso di un incontrollato accesso di immigrati nel territorio dello Stato italiano. Quindi, mi rivolgo con la massima serenità alla vostra valutazione che - sono certo - verrà presa nell'interesse dell'Italia, nel rispetto dello Stato e dei suoi poteri. Ricordo bene le parole con le quali ho giurato nel momento in cui ha assunto l'incarico di Ministro: ho giurato di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. È con questo spirito che ho agito sempre da Ministro dell'interno, nel rispetto dei miei doveri e della volontà del popolo sovrano.

Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'onore di potere Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'onore di potere difendere il mio Paese e i miei figli con il mio lavoro, che penso di svolgere con onestà, con buonsenso, con coraggio. Comunque votiate, io vi ringrazio e siate certi che continuerò fare questo mio lavoro senza nessuna paura, altrimenti farei un altro mestiere. Per l'Italia. Senatore Marcucci, lei conosce meglio di me il Regolamento, quindi non protesti per l'orario. Lo conosce meglio di me: posso stabilire fino a trenta minuti l'orario che ritengo, d'accordo? MARCUCCI Si tranquillizzino gli amici di sinistra che hanno sforato il loro tempo. Io risparmierò a quest'Assemblea e agli italiani due minuti perché vorrei semplicemente concludere che, amando l'Italia, amando i miei figli, amando i figli degli italiani, dedico la mia vita a questo splendido Paese. Grazie di cuore.

penso che sia necessaria una replica per ribadire le motivazioni di natura anche giuridica e costituzionale che hanno portato il relatore, con un voto largamente prevalente della Giunta, a proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere. Io ho ascoltato quasi tutti gli interventi dei colleghi e ho sentito motivazioni, per carità, interessanti, ma molte volte di natura politica. Mi sono anche reso conto - e non è colpa di nessuno - che non tutti hanno letto le sedici pagine di atto parlamentare della relazione

(penso alla senatrice Malpezzi), che hanno apprezzato il metodo seguito. Poi, sul merito, le opinioni sono diverse. In molti casi però ho visto che dei colleghi hanno fatto delle affermazioni di natura politica legittime. Io stesso ieri, quando si parlava della Cina, ho svolto una dichiarazione di voto per il mio Gruppo, molto polemico nei confronti del Governo. Poi, dopo pochi minuti, da relatore e Presidente della Giunta, ho svolto un intervento in base alla funzione che ho avuto l'onore di svolgere in questa legislatura e sulla base del diritto e delle leggi vigenti. Altri colleghi non condividono la politica di Governo? Hanno le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni di sfiducia. Il Regolamento consente a ciascuno di noi di esercitare in altri ambiti la critica politica. Qui stiamo parlando di una vicenda che è stata incardinata secondo le regole. Voglio dire, nella mia replica, che alcuni hanno fatto anche confusione, l'articolo 51 del codice penale qui non è in questione. Recita l'articolo 51 del codice penale: «L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità». Qui non siamo in questo caso. Qui siamo - l'ha ricordato prima con precisione il presidente Casini - di fronte all'applicazione della legge costituzionale n. 1 del 1989, perché un *referendum* nel 1987 ha abolito la Commissione inquirente e i membri del Governo sono stati affidati alla magistratura ordinaria. La citata legge del 1989 regola questa procedura dando all'Assemblea di appartenenza - ed è questo il caso in cui ci troviamo - la possibilità di valutare se sussistano o no quei requisiti quei requisiti dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale del 1989, e che ci siano delle esimenti, cioè non si concede l'autorizzazione a procedere al processo se - una «tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» o «il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Io ho sentito affermare, nelle relazioni di minoranza e negli interventi, cose che non ritengo siano vere. Ieri, la senatrice Bonino - la cito per l'autorevolezza e per l'anzianità di mandato - ha detto che io non ho motivato nella relazione il preminente interesse pubblico. Le ho mandato una copia della relazione, che evidentemente non aveva letto, perché non solo io ho spiegato, in questo caso, dove si ravvisa il preminente interesse pubblico, ma ho anche spiegato che non c'è - colleghi che parlate di impunibilità totale - la possibilità, in base a questa legge, di dar luogo a una impunità assoluta per i membri del Governo. Ho fatto anche degli esempi: se un membro del Governo prende dei soldi perché autorizza un'opera pubblica, non ci può essere nessun preminente interesse pubblico; se ci sono lesioni irreversibili di diritti della persona o una persona dovesse morire, non c'è possibilità di tutelare un'azione di Governo, perché lesioni irreversibili meriterebbero un processo e il soddisfacimento di interessi privati non meriterebbe il rango di tutela dell'interesse pubblico. Leggete la relazione! Votate contro, ma non negate la verità dei fatti e le motivazioni che sono state scritte con precisione e dovizia di particolari. Abbiamo fatto anche degli esempi *a contrario*, nella relazione: se non ci fosse stato un interesse pubblico nell'azione del ministro senatore Salvini, quale sarebbe stato l'interesse privato nel caso specifico? Ma se ci fosse stato un interesse politico-partitico, avrebbe agito per un interesse di parte: nella relazione, cari colleghi - lo dico a coloro che hanno svolto interventi critici - ho riportato interi brani dell'intervento che il presidente del Consiglio Conte ha svolto il 12 settembre in quest'Aula. A chi ha detto che non c'è la circolare condominiale, in cui il Governo ha scritto una lettera, ricordo che il Presidente Presidente del Consiglio è venuto a raccontare la sua condivisione dell'azione del Governo in quest'Aula. È un dato di fatto o no? Conterà qualcosa un intervento in sede parlamentare! Lo dico distinguendo i giudizi politici - anche i miei

Per favore, un attimo di attenzione, sta replicando il relatore. Per quanto riguarda poi le altre questioni dell'azione di Governo, il Presidente del Consiglio ha svolto un intervento, quindi l'interesse pubblico c'è: la trattativa con Malta, che non concedeva il POS, la trattativa con l'Unione europea, con le riunioni, gli ordini verbali ai rappresentanti che si sono recati il 24 agosto a Bruxelles, è tutto scritto nella relazione, quindi prescindo perfino dagli interventi dell'interessato e di altri, che pure hanno prodotto documenti che abbiamo letto. Abbiamo letto gli atti del Senato, in primo luogo, che ci hanno dato una traccia. Il Presidente del Consiglio, anche prima e dopo, era intervenuto sulle linee di politica dell'immigrazione del e quindi l'interesse pubblico, come scrivo nella relazione, è anche stato rappresentato dal tentativo di dare una regolamentazione più rigorosa e corretta della gestione dei flussi migratori. È un interesse pubblico, si può politicamente condividerlo o no. Non c'è un'esimente assoluta per qualsiasi comportamento e abbiamo motivato la sussistenza sussistenza delle esimenti. Crediamo quindi che la relazione possa essere assolutamente approvata dall'intera Assemblea, perché anche *a contrario* non ci sono interessi personali, non ci sono interessi partitici, perché gli interventi del Presidente del Consiglio ci sono stati. Quanto alle preoccupazioni per l'ordine e la sicurezza, nella relazione viene citato ciò che,

al Parlamento dei Servizi segreti. Io non so se i Servizi segreti vaneggino, ma se fossi Ministro mi preoccuperei delle relazioni dei Servizi segreti rese al Governo e al Parlamento. Si potrebbero dire molte altre cose, ma non voglio sforare il tempo, caro Presidente. Dagli interventi non ho colto argomenti che abbiano indotto il relatore a cambiare idea o a cambiare relazione. Si è parlato di bilanciamento dei diritti, delle esigenze di preminente interesse pubblico. Mi dispiace che la senatrice Bonino non ci sia, starà leggendo la relazione che le ho dato ieri, perché ha detto che non avevo motivato: imparare a leggere è doveroso, perché si può non essere d'accordo, ma non negare l'evidenza. Noi abbiamo fatto un lavoro in Giunta e voglio ringraziarne tutti i membri, comunque la pensino, perché abbiamo approfondito la questione. Non creiamo un precedente:

se mai dovesse accadere, ora o in futuro, ma abbiamo riportato anche gli esempi *a contrario*: abbiamo scritto i casi in cui non si potrebbe mai concedere un'autorizzazione, perché sappiamo che il lavoro che il Senato sta facendo in queste settimane e che la Giunta ha fatto ha una sua rilevanza. Non ci sono precedenti recenti di così grave rilevanza, quindi abbiamo scritto e soppesato parole e atti affinché non dovessero creare equivoci e potessero essere utilmente

96 della Costituzione, e il relatore ha offerto motivazioni a quest'Assemblea, che spero saranno condivise. Auspico, quindi, che venga approvata la relazione che ho proposto, per negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro senatore Salvini.

Non v'è dubbio che il ministro Salvini abbia deliberatamente operato la scelta di perseguire gli obiettivi del Governo in spregio dei diritti dei 177 naufraghi a bordo della Diciotti: più ministeriale di così!

Era necessario questo sacrificio in nome di un preminente, insopprimibile interesse pubblico? La risposta è no. Pur riconoscendo il più ampio grado di autonomia del Governo nella determinazione della propria azione e dei mezzi necessari per assolverla, è evidente che essa sia sempre e comunque subordinata al preminente interesse pubblico, che si sostanzia nel rispetto della Costituzione e dei suoi principi fondamentali. L'adesione concreta e quotidiana al dettato costituzionale rappresenta un obbligo giuridico, politico nonché morale di ogni cittadino e, in particolare, di chi serve le istituzioni. Nessuna delle tesi a difesa dell'operato del Ministro, a mio avviso, appare fondata. Ci ha detto che c'è un solo morto nel 2019.

La percentuale di morti è passata dal 3,4 per cento del 2018, all'11,5 per cento del 2019. Insomma, la traversata non è mai stata così pericolosa come oggi

problema con Malta. È vero che il comportamento di Malta è stato esecrabile sotto tutti i punti di vista e anche da un punto di vista morale, ma non si trattava di una controversia internazionale. Si trattava di far rispettare rispettare quello che il presidente Conte era riuscito a ottenere in una precedente riunione del Consiglio europeo, ovvero l'adesione volontaria nella redistribuzione dei migranti. Ciò emerge dagli Ciò emerge dagli atti, ma anche dalle ammissioni dello stesso ministro Salvini. L'ordine di non far sbarcare i naufraghi è stato emesso per esercitare una pressione nei confronti degli altri Stati dell'Unione europea, che avrebbero dovuto volontariamente assumersi la ripartizione dei migranti. È evidente quindi l'intento di strumentalizzare il caso Diciotti, ben prima dell'attracco a Catania, per ottenere in modo forzoso quella che doveva essere una volontaria adesione degli altri Paesi dell'Unione europea. Il tentativo di superare il Regolamento di Dublino a favore di politiche che prevedono logiche diverse di distribuzione a livello europeo dei migranti è certamente condivisibile e legittimo, ne siamo perfettamente consapevoli e sposiamo integralmente questa politica a livello europeo. Fare pressione politica sull'Europa o, più correttamente, coazione morale, al fine di cambiare i regolamenti - perché è il Regolamento di Dublino che dovete cercare di cambiare a livello europeo trattenendo esseri umani a bordo di una nave italiana, è invece del tutto illegittimo. Altre tesi illustrate dal relatore non trovano la nostra condivisione. trova certamente quella secondo cui l'imbarcazione possa essere considerata come luogo sicuro, perché sono stati sequestrati dei naufraghi oltre il tempo strettamente necessario per procedere allo sbarco sulla terraferma, dove deve completarsi la procedura di salvataggio in mare. mare. Questa è un'evidente violazione delle convenzioni internazionali, che costituiscono norme di rango primario e di rilevante interesse costituzionale, in virtù degli articoli 2, 10, 11 e 117 della Costituzione.

nemmeno accoglibile la tesi che vede nella libera circolazione, invece che nella libertà personale, il diritto compresso. La libertà personale è solennemente riconosciuta e protetta dall'articolo 13 della Costituzione; la libertà di circolazione è ugualmente prevista dall'articolo 16 della Costituzione e nessuna prova dei motivi di sanità e di sicurezza che l'avrebbero potuta limitare è stata prodotta. prodotta. La nostra Costituzione prevede anche che «Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche» mentre è stato proprio il Ministro a motivare la sua azione con ragioni politiche, ponendosi quindi, di fatto, anche volendo assumere la tesi della compressione della libertà di circolazione, al di fuori dell'articolo 16 della Costituzione. È dunque palese come anche nella ricostruzione del relatore vi sia una totale confusione tra il diritto all'immediato sbarco dei naufraghi e le obbligatorie procedure di identificazione, ovvero una fase successiva, concernente la gestione a terra dei migranti. Essi diventano migranti, ma prima sono naufraghi che devono sbarcare. Quelle del ministro Salvini appaiono anche giustificazioni deboli, al punto che, nemmeno nella prima parte della sua relazione, il relatore ha ritenuto di tenerne conto.

per esempio, tra la baldanza con cui ha aperto le comunicazioni giudiziarie del tribunale, in diretta su Facebook, e la compostezza giuridica della lettera al «Corriere della sera», con cui, con una sorprendente giravolta, è passato dal «processatemi pure» al «chiedo al Senato di salvarmi dal processo». Ulteriori giustificazioni riguardano la tutela dell'ordine pubblico e la difesa dei confini, ma basta ricordare che i naufraghi erano già in territorio italiano. Signor Ministro, l'articolo 4 del codice penale stabilisce che le navi italiane sono considerate vale, incontrovertibilmente, per ogni imbarcazione battente bandiera italiana, figuriamoci per una nave militare come la l'ordine pubblico delle persone inermi, fortemente provate da giorni e giorni di navigazione, in fuga da guerre, stupri e violenze,

Si è detto poi che c'erano infiltrazioni di tipo terroristico. Pur condividendo la preoccupazione in via generale, non si può non rilevare che nel caso specifico si trattava di 177 naufraghi in custodia delle autorità autorità italiane, quasi totalmente provenienti dall'Eritrea, cioè da un Paese per il quale si prefigura l'accoglimento di eventuale richieste di protezione internazionale. Né l'autorità giudiziaria, né gli organi competenti antiterrorismo, né i servizi segreti che sono stati evocati hanno ravvisato un pericolo concreto di infiltrazione terroristica sulla persone sono state tutte identificate già a bordo e i dati sono stati trasmessi dalla procura di Agrigento agli organi polizia e non è stato rilevato alcunché addirittura nella fase Davvero si vuole giustificare il sequestro con questa motivazione? E allora perché i naufraghi, poco dopo lo sbarco, sono potuti fuggire? Abbiamo affidato a Paesi che si erano offerti per l'accoglienza dei probabili terroristi?

le argomentazioni del relatore in merito alla valenza governativa del cosiddetto caso Diciotti sono in aperto contrasto con la memoria difensiva. Il presidente Gasparri ha spostato l'intera titolarità delle azioni e delle politiche del Governo sul presidente del Consiglio Conte, ma sappiamo che ogni Ministro è individualmente responsabile degli atti del proprio Dicastero.

quale preminente interesse pubblico non si sarebbe tutelato se i 177 naufraghi fossero sbarcati e avessero atteso, presso gli *hotspot*, la decisione degli altri Paesi dell'Unione europea circa la volontaria accoglienza dei migranti? Non abbiamo avuto risposta. Potevano stare a terra e non restare nella nave.

ha stabilito che compiere azioni dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica e la libertà personale non è consentito nemmeno in nome del supremo interesse pubblico cui ci si sta muovendo è dunque molto pericoloso. Per questi motivi, il Ministro non si dovrebbe sottrarre al giudizio della magistratura (si badi bene: al giudizio, non alla condanna).

ed è questo e solo questo che ci deve interessare qui, non altro. Qui dobbiamo occuparci di una domanda specifica che ci pone la magistratura: il tribunale dei Ministri di Catania; non dobbiamo occuparci di altro. Il perimetro del nostro discorso è molto importante, perché altrimenti la nostra espressione potrebbe essere sindacata da altre istituzioni. Il nostro è un giudizio insindacabile, sempre che sia coerente, non contraddittorio e pertinente. questo è importante verificare che la decisione di bloccare la catena di comando che doveva condurre all'obbligatoria indicazione del POS è evidente responsabilità del ministro Salvini per sua stessa ammissione, così come - ancor più chiaramente - l'adozione del divieto di sbarco, il quale ha compresso in maniera chiara e illecita, secondo il tribunale, la libertà personale dei naufraghi, che sono stati trattenuti senza motivo sulla nave

si sarebbe potuto procedere con ordine alla loro identificazione e a raccogliere le loro eventuali richieste e nulla di tutto quello di cui oggi stiamo discutendo sarebbe successo. È stata una violenza del tutto gratuita. Per giustificare la scelta del Ministro e le sue conseguenze la relazione della maggioranza si avventura in teorizzazioni discutibili e ritiene impossibile che vi possa essere un reato ministeriale allorquando si sia di fronte ad una lesione irreversibile dei diritti fondamentali; sempre secondo la relazione, si sarebbe di fronte ad una lesione irreversibile dei diritti fondamentali allorquando l'ipotetica lesione dei diritti colpiti è così grave da alterare la natura stessa del reato. fa quindi? Si crea una gerarchia di diritti fondamentali che non esiste; crea una gerarchia dei diritti fondamentali tra la vita, la salute e la libertà personale, come se la libertà personale non fosse anche la libertà morale, non fosse anche una libertà comprensiva che pertiene alla vita.

con questo modo di ragionare - forse è stato già accennato - non potremo punire alcuna ipotesi di sequestro che abbia per così dire il buon fine, magari dietro pagamento del riscatto. del riscatto. È semplicemente una sciocchezza. Il diritto alla vita non va infatti inteso come diritto alla vita biologica, ma come diritto alla libertà della persona in senso pieno.

che ponga essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi...». tale speciale causa di giustificazione «non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita,

sussistere una valida ragione; nemmeno la sicurezza nazionale è dunque ipotizzabile come valida ragione per derogare ai diritti inviolabili della persona.

lo Stato e quindi anche il legislatore nazionale. La citata risoluzione ha come scopo come scopo il fatto di alleviare il comandante della nave dai propri obblighi corrispondentemente agli obblighi del Governo contraente di coordinamento e cooperazione

La parte che viene citata, a sproposito, dal collega Pillon si trova al punto 6.14 di questa risoluzione.

che una nave in assistenza non dovrebbe essere considerata un *place of safety.* Anche

non soltanto richiamandoli alla loro battaglia di principio per l'abolizione della prerogativa dell'immunità, ma perché in questo caso non si tratta di applicare una prerogativa funzionale: si tratta di un odioso privilegio si tratta di un odioso privilegio svincolato da qualsiasi criterio obiettivo. Per questo

ricordare, tra l'altro, che si sta votando una relazione che nei criteri di giudizio non è per niente dissimile da quella del 13 febbraio scorso, nella quale si leggeva che non esisterebbe

«Si osserva a tal proposito che l'autonomia della funzione di governo presuppone anche un'autonomia nella scelta dei mezzi e non solo quindi dei fini da perseguire». In pratica, veniva evocato un machiavellismo pericoloso che avrebbe consentito l'uso di qualunque mezzo il Governo ritenesse utile per raggiungere un fine da esso stesso prefissato. Concludo e spero anche di aver ottenuto un minimo d'ascolto da parte dei miei colleghi del MoVimento 5 Stelle. come tutti i cittadini, anche i Ministri, se nell'esercizio delle loro funzioni commettono dei reati, devono risponderne davanti alla giustizia, quali che siano le motivazioni politiche a fondamento delle loro azioni. L'unico caso in cui è possibile evitare il processo è che il Parlamento, con giudizio insindacabile, ritenga di non concedere l'autorizzazione a procedere. Vale per tutti i Ministri di qualsiasi Governo, attuale e futuro: occorre tenerlo bene a mente. In questo caso il diniego dell'autorizzazione a procedere aprirebbe a pericolose derive autoritarie, per evitare le quali

Se qualunque Ministro fosse autorizzato a violare impunemente la legge con atti di natura politica, senza che la magistratura potesse sottoporlo a giudizio, si darebbe luogo ad un pericoloso precedente: il rischio sarebbe quello di fornire, in futuro, una giustificazione a qualunque crimine in nome di un fine politico. Il delicato compito del Senato attiene squisitamente a un giudizio sui mezzi usati e sui fini che si volevano perseguire; a un saggio e approfondito contemperamento tra i beni protetti dalle norme violate e i mezzi usati dal Ministro per attuare la politica del suo Governo. Il ministro Salvini ha certamente posto in essere un comportamento in violazione delle norme internazionali e nazionali e ha, secondo il tribunale dei Ministri di Catania, abusato delle funzioni attribuite al Ministro dell'interno al Ministro dell'interno ponendo arbitrariamente il proprio veto all'indicazione del POS, determinando cosi la permanenza forzosa dei naufraghi a bordo della nave Diciotti, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile e certamente al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Le ragioni che hanno determinato il sequestro esulano da valutazioni di tipo tecnico. L'ordine è stato infatti dato per ragioni connesse alle trattative in corso in sede europea:

Un grande Paese non usa come ostaggi per una trattativa internazionale una nave militare, il suo equipaggio e i naufraghi salvati. Non c'è alcun dubbio che il comportamento di Malta sia stato esecrabile ma non risulta che l'Italia abbia sollevato, nelle sedi opportune, alcuna controversia internazionale. Non c'è alcun dubbio che la sicurezza del Paese debba essere una priorità, ma nel caso specifico non risulta alcuna minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza, come dimostra il fatto che nessun provvedimento amministrativo o giudiziario sia stato emesso nei confronti dei naufraghi, una volta scesi a terra. Quale emergenza, quale catastrofe si sarebbe abbattuta sul nostro Paese? Quale preminente interesse pubblico non si sarebbe tutelato se i 177 naufraghi fossero sbarcati e avessero atteso presso gli *hot spot* le decisioni degli altri Paesi dell'Unione europea? Quale articolo della Costituzione autorizzava il ministro Salvini a impedire lo sbarco? Nessuno. La Costituzione, al contrario, agli articoli 2 e 10, difende i diritti fondamentali irrinunciabili così come quello della libertà personale. Non vi è dubbio che il Ministro abbia agito al di fuori delle finalità proprie dell'esercizio del potere conferitogli dalla legge in quanto le scelte politiche non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati di garantire, nel modo più sollecito, il soccorso e lo sbarco dei naufraghi in un luogo sicuro, obblighi che derivano da convenzioni internazionali e costituiscono una precisa limitazione alla potestà legislativa dello Stato in base agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione. Anche le sentenze della Corte costituzionale hanno evidenziato come la discrezionalità politica nella gestione dei fenomeni migratori non possa mai entrare in contrasto con la Costituzione e con i trattati internazionali. Ne consegue che la decisione del Ministro non trova alcuna giustificazione ma anzi contrasta apertamente con la tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti. Ogni espressione di indirizzo politico e di governo non può, infatti, avere capacità lesiva di situazioni soggettive individuali, dovendo sottostare al principio supremo di legalità e avendo il suo contrappeso principe nella Costituzione e nei diritti inviolabili in essa indicati, tra cui spicca - lo ripeto ancora una volta - il diritto alla libertà personale. Il preminente interesse pubblico è in qualche modo assimilabile al concetto di ragion di Stato, che trova però, giustamente, il suo limite nella garanzia dei diritti inviolabili della persona umana. Su questo aspetto, come ho già illustrato, è illuminante l'articolo 17 della legge n. 124 del 2007 sui servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica. Secondo tale articolo non può essere autorizzata né giustificata la condotta prevista dalla legge come un reato diretto a mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica e la libertà personale di una o più persone, neanche per la difesa della sicurezza nazionale. Gli obiettivi del contrasto al traffico di esseri umani e della condivisione della responsabilità con gli altri Paesi europei sono legittimi ma non sfuggirà che ciò che rileva in questa sede è solo la modalità attraverso la quale il Ministro dell'interno abbia inteso realizzarli. Qualora egli avesse voluto sollevare il tema dell'equa ripartizione dei migranti in ciascun Paese europeo, avrebbe potuto e dovuto farlo nelle sedi opportune, dopo averli fatti sbarcare, così come prevedono le convenzioni internazionali. L'individuazione del POS è affidata al Ministero dell'interno e non al Governo. L'omissione di quell'atto è stata una precisa responsabilità personale del Ministro. A nulla, se non a giustificare all'esterno il voto di oggi, rilevano le successive prese di posizione del presidente Conte e dei ministri Di Maio e Toninelli. i fatti e i comportamenti del ministro Salvini sono stati valutati da più magistrati (è stato detto anche dallo stesso ministro Salvini). Il tribunale dei ministri di Catania ha ritenuto di individuare un'ipotesi di reato e correttamente si è fermato, rivolgendosi al Senato. Sta a noi, dunque, decidere non se il Ministro sia colpevole o innocente ma se debba o no essere sottoposto al giudizio della magistratura. Bisogna quindi concentrarsi su due profili: il primo è quello della rilevanza, il secondo quello della preminenza. Il legislatore costituzionale sembra, con questi aggettivi, suggerire che il bilanciamento dei valori in gioco, ai fini della concessione o del diniego dell'autorizzazione, debba risolversi a favore della tutela dei più alti valori del nostro Stato. E quali sono i più alti valori della nostra Carta costituzionale, se non il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo? Sovvertire l'ordine, dare priorità ad altri interessi rispetto ai diritti inviolabili, quali quello della vita e della libertà costituzionalmente protetti, significherebbe ammettere una nuova, ma pericolosa, concezione della ragion di Stato. I diritti fondamentali non devono mai essere compressi per esigenze politiche. Trattenere delle persone in un luogo senza un atto motivato dell'autorità giudiziaria configura un reato, che deve essere sottoposto al giudizio della magistratura. Votando contro l'autorizzazione a procedere si crea un grave e pericoloso precedente, che mina nel profondo il senso stesso della nostra democrazia e il suo complesso ma equilibrato sistema di pesi e contrappesi, di tutela dei diritti inviolabili della persona. Piegando la Costituzione alle esigenze contingenti di questo Governo, noi ci apprestiamo a cancellare secoli di diritto e oltre settant'anni di storia repubblicana. Vale oggi per i naufraghi della Diciotti, ma domani potrà valere per chiunque. il diritto e coi diritti fondamentali non si scherza. Le convenienze politiche del momento, magari nascoste dietro il voto di una manciata di sostenitori attraverso una piattaforma *web* privata, non possono sottomettere la cultura giuridica e la tutela della Costituzione ad interessi di parte. Nessuno si stupisca se, da cittadino, mi auguro che il Ministro dell'interno della Repubblica italiana sia ritenuto innocente rispetto al reato a lui contestato.

Pertanto, si propone la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 89.

l'intervento del ministro Salvini, preceduto dalla replica del Presidente della Giunta, rendono superfluo affrontare dal punto di vista tecnico, giuridico e anche umano la questione. Ho pensato allora di cambiare completamente il mio intervento e di cercare di fare quello che correttamente, e credo, intelligentemente, non ha fatto il ministro Salvini. Risponderò, cioè, alle obiezioni

di una vicenda strettamente politica, ma meno adatto a una vicenda in cui invece il Parlamento e, in particolare, il Senato è chiamato a svolgere una funzione giurisdizionale. La

dal processo». Ma il processo è qui, cari colleghi: la legge attribuisce oggi al Senato un compito giurisdizionale. Ci attribuisce il compito di decidere se c'è o non c'è l'interesse pubblico preminente nell'esercizio dell'azione di Governo in ciò che ha commesso Salvini per conto di tutto il Governo, come si evince abbondantemente dalle parole del Presidente del Consiglio in quest'Aula - non le ripeterò - che costituiscono certamente linea di indirizzo governativo.

che questo è uno scontro tra chi sostiene il Governo e chi non vuole il Governo: sbagliato. Noi non siamo maggioranza, noi non sosteniamo il Governo. Se dovessimo attenerci al *cui prodest*, ci servirebbe allora moltissimo creare zizzania, vedere mandato a giudizio Salvini e far saltare il Governo, che è uno degli obiettivi

questi diritti sono stati compressi troppo a lungo e non abbiamo visto processi nei confronti di chi ha consentito con la propria inerzia e con la propria azione politica

E allora dov'è questa violazione, se anche non ci fosse il preminente interesse? Dov'è? Una volta sbarcati voi avete la riserva mentale di sapere che sarebbero stati liberi, come lo sono stati, perché quelli sbarcati poi sono scappati La verità è che

a maggioranza in tale sede, è la strenua difesa della posizione del tribunale dei Ministri; ha ragione la magistratura, ci dobbiamo inchinare alla magistratura. Che cosa Zuccaro? Un esponente di Fratelli d'Italia? Zuccaro è un esponente della Lega? Un esponente del MoVimento 5 Stelle? Zuccaro è un pubblico ministero, un uomo probo,

ha sempre avuto un amore sviscerato per i pubblici ministeri e meno per i giudicanti. Se solo Zuccaro avesse detto il contrario e il tribunale dei Ministri avesse invece preso la sua posizione, oggi

vicende. Il Consiglio europeo del 28 giugno ha raccomandato - testualmente - che per smantellare il traffico di esseri umani ed evitare la tragica perdita di vite umane è necessario eliminare ogni incentivo a intraprendere viaggi pericolosi. Se dovessi svolgere un intervento solo politico, direi che questa è la critica che faccio al Governo: ci vuole il blocco navale, non dobbiamo proprio farli partire, così eliminiamo il problema dello sbarco o del mancato sbarco. Le parole del Consiglio europeo testimoniano esse stesse che vi è un interesse certo da parte dello Stato a controllare i flussi migratori. Non si tratta di un diritto inviolabile; non è un diritto inviolabile quello di poter entrare liberamente nel nostro Paese, nella nostra Patria, nella nostra casa. *(Applausi dal sancito dalla Costituzione; al contrario, è vietato! Un Governo che si preoccupa di di controllare chi entra e chi non entra a casa nostra è un Governo che fa il suo dovere. Voi volete processare Salvini perché ha fatto il suo dovere. Questa è la verità. Certo, io capisco, ci sono due visioni culturali opposte: una è aperta a qualunque arrivo, all'assenza di controllo di ogni flusso migratorio perché dice che è inevitabile - ed è vero

accollasse il compito di aiutarci già ne avremmo di meno. Tuttavia, ammesso che sia inevitabile, ciò non vuol dire che da parte dei Governi sovrani non ci debba essere una pratica normativa, legislativa e di sicurezza tesa a controllare e a gestire questi flussi. Ecco il preminente interesse. Concludo, e ringrazio il Presidente se mi dà qualche secondo ancora, con una notazione leggera: c'è un film che tutti forse abbiamo visto. È un film con Tom Hanks, Terminal» - ve lo ricordate? - in cui un cittadino di un Paese imprecisato rimane all'interno di un terminal aeroportuale; non può tornare indietro, come i nostri migranti, perché nel suo c'era la rivoluzione; non può sbarcare perché non ha le carte in regola. quindi lasciato per mesi nel terminal senza neanche assistenza, senza neanche cure sanitarie. Vogliamo imputare il Governo americano - in un caso del genere - di violazione dei diritti umani? Non ci ha pensato nessuno. Voi ci avreste pensato.

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi, ringrazio il Ministro per aver accolto l'invito a essere presente in Aula in un momento così importante per la storia repubblicana e per la storia della democrazia parlamentare. Signor Ministro, oggi lei ci ha parlato d'altro, non della vicenda di cui dobbiamo discutere. Ci ha parlato del suo amor patrio - condividiamo e apprezziamo - così come dell'amore per la famiglia

sul numero degli aumenti degli sbarchi con altri mezzi che le ha proposto il collega Mirabelli. Oggi noi discutiamo di una cosa molto precisa, inconfutabile. Non dobbiamo discutere se aveva ragione Malta o su come si è comportata Malta. Il punto del discrimine - attenzione - l'ha segnato il tribunale di Palermo, ossia il tribunale che voi spesso citate per evocare un'archiviazione che nel merito non c'è stata. Il tribunale di Palermo ha stabilito molto chiaramente quando

che ha delineato quali sono le condotte rilevanti a partire dalle quali è da considerare valida la richiesta di POS e l'inizio di una procedura; a partire dalle quali non ha assolutamente più rilevanza se Malta doveva farsi carico o no; a partire dalle quali è l'Italia, nel momento in cui soccorre, che ha l'onere e l'incarico di portare a compimento un'operazione di soccorso. Operazione che comprende non soltanto il prestare delle cure - e ci mancherebbe altro -, non soltanto sfamare - e ci mancherebbe altro - , ma comprende l'individuazione di un porto sicuro, lo sbarco e lo sbarco e comprende - sicuramente non viene eluso o sostituito dalle operazioni a bordo - l'identificazione e il portare a termine tutti gli adempimenti. Tutto questo incombe sullo incombe sullo Stato italiano, che è tale a partire dalla nave Diciotti. Quali confini? La nave Diciotti è già Stato italiano. Stato italiano. Quale protezione per 177 persone, di cui ventisette minorenni e undici donne che avevano subito violenza sessuale? Di questo stiamo discutendo e questa è la dinamica temporale. è che sono state tenute in ostaggio per diversi giorni ben 177 persone e oggi, tra un amor patrio, una commozione familiare, lei, signor Ministro, ci ha ricordato che quei quattro giorni leggasi privazione della libertà personale garantita con doppia riserva di legge della Costituzione, ossia riserva di provvedimento e e ordine dell'autorità giudiziaria, per privare, ai sensi dell'articolo 13, un cittadino di qualsiasi nazionalità della libertà personale - sono serviti a svegliare qualcuno con cui si stava trattando. Questo è il paragone. Il reato ipotizzato, il sequestro di persona, è servito per svegliare qualcuno.

che una minaccia terroristica anche per i Servizi segreti comporta l'obbligo, se circostanziata, di riferire immediatamente all'autorità giudiziaria; e deve essere immediata e circostanziata. Non ci venite a parlare di una generica minaccia terroristica, che peraltro, se fosse stata seria, avrebbe dovuto imporre una sorveglianza particolarmente attenta anche quando gli immigrati sono sbarcati. Viceversa, questo, come sappiamo, non è assolutamente successo. PD)*. E allora di cosa stiamo discutendo? Guardate, la relazione del presidente Gasparri ha sgomberato il campo da ogni e ci indica con grande chiarezza di cosa stiamo discutendo. Noi stiamo discutendo e decidendo se un mezzo scelto per esercitare una pressione sulle istituzioni europee al fine di indurle a concordare piani o solamente come pressione, possa essere non soltanto la violazione palese di una disposizione di legge,

senatore Gasparri. Presidente Gasparri, lei ha ragione, sarà un caso molto importante; non so se farà giurisprudenza, ma certamente costituirà uno spartiacque, perché è la prima volta che noi non discutiamo se vi sia una questione privata o una questione pubblica, ma discutiamo per la prima volta in queste Aule se il potere politico possa dirsi al di sopra della legge. Stiamo discutendo se possa violare la Carta costituzionale nei diritti fondamentali. È un salto È un salto che non c'è mai stato in quest'Aula. Io non so se sarà un precedente, ma certamente sarà un momento importante per la nostra democrazia. Il punto è che è stato sempre rivendicato con una diversa spavalderia e una diversa animosità da quella che oggi ci ha testimoniato il Ministro in Aula e non ha avuto il coraggio, signor Ministro, di essere così chiaro e diretto come è stato il presidente Gasparri quando ha rivendicato questo potere, questa concezione dello Stato.

La seconda è che non c'è stata alcuna necessità o attività di difesa dei confini: erano già sul territorio italiano e c'era un dovere stabilito per legge di portare a termine una procedura. Non c'è alcuna attività o decisione o decisione di Governo che possa esimere o far diventare un interesse pubblico qualcosa che non lo può essere. In primo luogo, non c'è stato alcun Consiglio dei Ministri, in secondo luogo, le cronache dell'epoca testimoniano che c'era una dialettica molto aspra all'interno del Governo. Il ministro Salvini ha minacciato di dimettersi e il Presidente del Consiglio Conte era impegnato in modo instancabile a dissuaderlo dal persistere in quella condotta. Giustificare posteriormente, con una politica sui flussi migratori, è assolutamente inconferente. E giustamente il Presidente del Consiglio, essendo anche un avvocato, si è guardato bene dal rivendicare la legittimità del mezzo, che è esattamente l'unica cosa di cui noi stiamo discutendo. Vorrei anche sgomberare il campo dalla *fake* del coraggio e dell'eroico capitano a tutela di tutti noi (e arrivo alle conclusioni).

era stato assegnato il codice rosa, forse oggi il codice rosso, ma forse no, perché forse allora il codice rosso non sarebbe stato applicato. Voglio concludere, Presidente, che in quest'Aula - occasionalmente capita - il primo discorso della democrazia repubblicana di una donna in Parlamento sia stato fatto da Lina Merlin. Fu un discorso importante e toccante a difesa e per denunciare l'uccisione di un bracciante in uno sciopero nel Polesine. Fu un discorso a difesa della libertà, contro l'arbitro del potere. A questo ci richiamiamo e ci appelliamo. Perché qui, signor Presidente, non è in discussione un programma o non programma di Governo sulle politiche migratorie;

La libertà non è un concetto estraneo a nessuno in quest'Assemblea.

La legalità è il potere dei senza potere.

parlare. Il Partito Democratico voterà contro la relazione del presidente Gasparri, a difesa della della libertà di tutti i cittadini; quella libertà stabilita dalla Costituzione, che non può essere violata da nessuna maggioranza e nemmeno da un Ministro, benché animato d'amor patrio.

onorevoli colleghi, signor Ministro, cercherò di essere breve ma di riportare il dibattito al tema. Ho ascoltato tutti gli interventi, sia in discussione generale che in dichiarazione di voto. Devo dire che le norme di legge che sottendono la questione di cui ci stiamo occupando sono state interpretate in modi molto, ma molto diversi dalla loro interpretazione autentica ed è ciò su cui oggi noi siamo chiamati a decidere. Il tribunale di Catania, con la relazione del 7 dicembre 2018, ha chiesto al Senato il rilascio dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini in ordine al reato di sequestro di persona aggravato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è pronunciata per l'accoglimento della proposta formulata dal relatore, nel senso del diniego della richiesta di autorizzazione a procedere, attesa la sussistenza, nel caso di specie, dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico, nell'esercizio delle funzioni di Governo, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. Questo è il campo di azione su cui deve essere chiamato a pronunciarsi il Senato. In base a questa norma, il Senato è chiamato a stabilire in particolare se il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico, nell'esercizio della funzione di Governo.

del senatore Mirabelli)*. Questi sono gli atti ed è veramente difficile comprendere, per chi è abituato a frequentare le aule giudiziarie da un punto di vista professionale, come nessuno abbia fatto riferimento a questa circostanza, che non è né secondaria, né di poca importanza, perché attiene al merito della questione, quel merito di cui non dobbiamo certamente occuparci, ma che già il procuratore della Repubblica ha definito in termini di infondatezza della notizia di reato. Questo è scritto nella relazione del Tribunale di Catania-sezione reati ministeriali, a pagina 2, che ha escluso di dover valutare i risvolti politici che hanno determinato la decisione di impedire lo sbarco dei migranti e di dover verificare le motivazioni che hanno indotto il Ministro ad agire, nonché il rapporto che può sussistere tra il supposto reato e l'interesse pubblico della funzione esercitata. Ciò perché questi caratteri, secondo il tribunale dei ministri, non sarebbero comunque tali da giustificare obiettivamente il reato ministeriale nella sua consistenza giuridica, ma potrebbero solo eventualmente fondare il diniego di procedibilità. Questo è il tema che ci occupa. Non intendo entrare nel merito di siffatta impostazione e della distinzione proposta, perché in questa sede ciò è del tutto irrilevante. Infatti il Senato può negare l'autorizzazione a procedere non solo quando dubita della configurabilità del reato (e questo ce l'ha detto chiaramente lo stesso procuratore della Repubblica), ma anche quando, più semplicemente, senza esprimersi sulla sussistenza dei suoi estremi, ritenga comunque che ricorra una delle ipotesi di cosiddetta giustificazione politica menzionata nell'articolo 9. Quindi, per le stesse ragioni, neppure mi attardo ad osservare che dal punto di vista giuridico probabilmente il diritto di libertà personale, che secondo l'accusa sarebbe stato compresso illegittimamente con il trattenimento dei migranti sulla nave anche in caso di autorizzazione allo sbarco avrebbe subito condizionamenti e limiti, sulla base delle stesse leggi vigenti. Questa è una circostanza lapalissiana ed è riportata anche nella normativa di carattere internazionale ed europeo: i migranti, comunque, anche una volta sbarcati, come nel caso di specie, vengono poi trattenuti nei centri di identificazione e questa non è una limitazione della libertà personale, ma addirittura è un dovere imposto dalle norme. Conta qui, più semplicemente, stabilire se il fatto che viene contestato al ministro Salvini si inserisca in una precisa direttiva politica del Governo, peraltro condivisa da tutti i suoi

ma qui non può negarsi un'evidenza assoluta della condivisione del Governo sull'azione, che ha riguardato la nave Diciotti. Successivamente conta valutare se l'attuazione di questa direttiva politica condivisa vada considerata di interesse preminente rispetto all'eventuale tutela di diritti, che potrebbero essere stati temporaneamente compressi con il fatto oggetto di contestazione. Il dibattito non coinvolge il merito di quella direttiva. Non dobbiamo neppure stabilire se quella direttiva politica sia giusta o sbagliata, corretta o inadeguata, poiché il diniego dell'autorizzazione a procedere non comprende l'approvazione e la conferma della direttiva. Siamo chiamati esclusivamente a valutare se, per avventura, il collegamento logico tra il fatto contestato (trattenimento dei migranti all'interno della nave Diciotti per quattro giorni, perché questo è il termine della contestazione) e quella direttiva debba considerarsi pretestuoso, arbitrario e illogico, oppure se - al contrario - abbia un oggettivo, congruo e plausibile fondamento. Questo è il senso dell'interpello che ci è demandato, volto alla protezione delle scelte politiche del Governo, a fronte di possibili censure o sbarramenti da parte della magistratura. il limite ed è questo l'oggetto su cui ci dobbiamo pronunciare. La risposta al quesito mi sembra allora del tutto ovvia. Quali che siano le opinioni sul merito della direttiva politica, che sicuramente noi tutti condividiamo, nessuno può negare lo stretto collegamento logico e congruente tra quella direttiva e la decisione di non far sbarcare i migranti sul suolo italiano. *(Applausi dal si è limitato a mettere in atto esattamente ciò che tutto il Governo aveva stabilito sul piano della strategia di contrasto al fenomeno delle migrazioni irregolari.

dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Dunque, rimane il secondo passaggio. Quella direttiva esprime un preminente interesse pubblico rispetto al bene che sarebbe stato compromesso dal fatto contestato? Anche su questo punto non c'è dubbio che, come ha già detto il tribunale, non dobbiamo stabilire se ricorra una causa di giustificazione con riguardo al reato,

che è salito a bordo della Diciotti ha controllato lo stato in cui si trovavano i migranti ancora a bordo della nave e non ha ritenuto che si stesse perpetrando un reato, altrimenti avrebbe avuto l'obbligo di impedirlo

Mi accingo a concludere. In proposito è importante tener conto che la legge qualifica come insindacabile la decisione che ci apprestiamo ad adottare. Ciò indica inequivocabilmente che la valutazione di preminenza non deve essere effettuata con parametri giuridici, dovendo invece attenere - ancora una volta - al profilo squisitamente politico,

farlo. Il compito che ci è rimesso è estremamente agevole. La cosiddetta giustificazione politica alla base del diniego di autorizzazione a procedere non solo non richiede che si giustifichi l'eventuale reato, escludendone l'illiceità, ma neppure - dall'altro lato - che si condivida e si giustifichi la scelta politica. In conclusione, la decisione di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini discende, in definitiva, dalla considerazione tranciante che, se consentissimo ai giudici di giudicare sull'ipotesi di reato, essi finirebbero per giudicare la scelta politica del Governo e questo, secondo la Costituzione, non si può fare. Per questi motivi noi voteremo a favore della proposta del relatore e della decisione della Giunta e, quindi, contro il diniego all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini.

contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. Personalmente, signor Ministro, sono convinto che lei non abbia commesso il reato previsto dall'articolo 605 del codice penale,

è stata un buco nell'acqua, perché si è rinviato tutto alla volontarietà delle ricollocazioni e, quindi, alla buona volontà di un'Europa che è stata e continua ad essere cinica, ingenerosa e pregiudizialmente chiusa ad ogni forma di solidarietà.

ci saremmo mossi in una dinamica politica diversa. Qui però siamo tenuti a valutare l'interesse superiore del Paese, che lei ha portato avanti e che ha assicurato.

Esiste uno stato di terrore che non possiamo, né dobbiamo ignorare. Allora, signor Presidente del Consiglio, signor Ministro dell'interno, l'Italia faccia sentire la propria voce nel consesso internazionale per una verifica dell'esistenza o meno dei diritti umani in tutto quel territorio. Non bastano soltanto i pattugliatori, non basta soltanto l'attenzione bilaterale: occorre alzare il tiro su quello che sta succedendo in quel territorio, dove tanti uomini e donne vengono massacrati e torturati e addirittura affidano a barconi, in mano ai trafficanti che voi giustamente contrastate, bambini e minori, minori, nella speranza di un futuro migliore. Questa è una realtà che dobbiamo contrastare e credo che il Governo italiano abbia il dovere di portare nella sessione internazionale dell'ONU più vicina questo tema, una verifica e un'ispezione.

un partito sostiene il dittatore Maduro, l'altro partito di maggioranza lo contrasta; ma lo abbiamo visto anche sugli F-35, nonché sull'approccio nei confronti dell'apertura alla Cina: dobbiamo essere invasi dal mercato cinese o cercheremo di invadere il mercato cinese? due posizioni dialetticamente contrapposte, dove non vi è chiarezza né questo Parlamento è stato messo in condizione di pronunciarsi su questi futuri patti. Per non parlare della TAV, su cui, signor Presidente del Consiglio, l'Italia sta veramente rischiando di perdere ogni forma di credibilità internazionale. Io ho apprezzato la sua mirabolante capacità giuridica oltre che politica nel risolvere in quel fine settimana una crisi che era dietro le porte, era dietro le porte, ma il problema della credibilità e del mantenimento degli accordi internazionali, che è la pietra miliare della credibilità di un Paese, è aperto: cosa ne faremo della TAV?

di *impeachment* e che incontra i *leader* dei *gilet* gialli che massacrano e mettono a fuoco la Francia, Parigi, per protesta nei confronti di una repubblica democraticamente esistente. Dunque, il tema che vorrei sottoporre al Presidente del Consiglio più che al ministro Salvini è il pericolo di non essere credibili e di pagare il prezzo di scelte politiche di carattere economico sbagliate, perché lo stallo sta avvenendo anche

e un'altra politica che vede la soluzione di questo problema con la crescita, con la spesa produttiva, quella che ci chiede l'Europa e che non le abbiamo assicurato; l'Europa che ci ha imposto addirittura clausole di salvaguardia per 23 miliardi anziché 13 perché non si fida di noi. noi. Ci accingiamo a verificare, signor Presidente del Consiglio, dei dati devastanti: abbiamo una produzione industriale crollata del 12 per cento, lo *spread* è passato da 120 a 240, la pressione fiscale aumenterà dello 0,4 per cento, il debito pubblico

un tipo di alleanza del genere, che poggia le basi su due visioni di sviluppo di società diverse, possa durare a lungo. Signor ministro Salvini, io ho vissuto l'esperienza del governo Prodi, che era legittimamente voluto dagli elettori e che aveva assemblato delle realtà partitiche diverse tra loro (si passava dal collega Turigliatto al collega Dini); quell'Esecutivo ha avuto vita breve, perché la politica ha fatto le sue scelte, cioè il sistema è andato in stallo e l'economia non cresceva. Io temo - e lo dico nell'interesse del Paese senza alcuna polemica personale - che questo Governo che poggia su un contratto e non su una coalizione, su un'alleanza omogenea, su una piattaforma di valori condivisi, possa rischiare di arrecare enormi danni al Paese. Lo dico in piena serenità, in piena coscienza, con piena responsabilità. il centrodestra è un valore, non una formula di Palazzo. È un'aggregazione storica e spontanea di un popolo che si è riconosciuto in una grande alleanza liberale e riformista, che pone l'individuo e non lo Stato al centro della società. Questa è la filosofia liberale di Forza Italia che ci ha sempre trasmesso Silvio Berlusconi e che ci infonde quotidianamente con il suo impegno e con la futura discesa in campo.

Eravamo assieme. I suoi Ministri lo hanno condiviso e ho fatto nomi e cognomi; ci abbiamo messo la faccia, perché siamo tolleranti, ma sappiamo essere rigorosi quando si deve contrastare la criminalità organizzata. Siamo liberali, riformisti e difensori di una giustizia giusta e veloce e abbiamo coniato l'articolo 111 della Costituzione con il nostro Marcello Pera responsabile della giustizia: quell'articolo 111, ministro Salvini e ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, che rischia di essere messo in discussione con l'entrata in vigore dell'abolizione della prescrizione, ove lei non sarà in grado - e non sarà certo colpa sua - di riformare la giustizia in dieci mesi, riforma della quale non vi è traccia alcuna nei lavori parlamentari.

non di convenienza, come quello che sarà espresso a breve da qualche suo alleato, ma di coerenza della nostra storia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Il nostro voto di coerenza è un voto che onora la nostra credibilità, passata, presente e futura.

Credo che, a prescindere da come oggi voteremo e da quello che ciascuno di noi pensa, è a tutti chiaro che in quest'Aula oggi si stia svolgendo un dibattito di importanza straordinaria che ha pochi precedenti nella storia parlamentare di questo Paese. Un dibattito in cui abbiamo di fronte a noi senatori, che rappresentiamo la sovranità popolare e il potere legislativo, il Governo, che rappresenta il potere esecutivo di questo Paese che è portato in quest'Aula da un altro potere, quello giudiziario, affinché tutti noi senatori possiamo valutare le sue azioni. Oggi in quest'Aula nessuno può dubitare del fatto che stiamo affrontando il cuore della democrazia e che la democrazia si sta confrontando con se stessa e con i propri limiti: dobbiamo averlo chiaro. Qualcuno prima di me ha detto che il Governo non è al di sopra della legge. È verissimo: il Governo, il Parlamento e anche la magistratura in questo caso si stanno muovendo nella cornice della legalità repubblicana, secondo l'articolo 96 della

a tutela di un preminente interesse pubblico o di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante. L'articolo 9, al comma 3, parla di preminente interesse pubblico perché (e qui siamo nel cuore del problema della democrazia) non qualsiasi azione di governo potrebbe essere legittima sempre, solo perché azione di governo. Le azioni di governo vanno valutate secondo l'interesse costituzionale o il preminente interesse pubblico, cioè attraverso un bilanciamento che le norme rimettono a noi senatori, in questo caso. Tale bilanciamento è con

dalle nostre Forze dell'ordine, dalla Marina e da tutto l'apparato dello Stato dentro un porto della Repubblica, al sicuro finalmente, per quattro giorni, prima, durante e dopo i quali l'intero Governo, come ha ricordato il Presidente del Consiglio nel primo intervento in quest'Aula a settembre, si era impegnato per una cosa che per noi del MoVimento 5 Stelle è importante da quando siamo in Parlamento. È dal 2014, infatti, che contestiamo i folli Trattati sottoscritti prima del nostro arrivo in Parlamento e che facevano sì che chi sbarcava in uno Stato diventasse e rimanesse problema di quello Stato e non sbarcasse in Europa. Noi abbiamo sempre detto, dal 2014, che chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Il Presidente Conte è andato a dire questo a giugno, prima che arrivasse la nave Diciotti in Europa,

ha perseguito, impedendo per quattro giorni lo sbarco dei migranti nel porto di Catania, sbarco che avrebbe determinato l'immediata applicazione di quei Trattati che noi contestiamo da sempre.

ma erano questioni vergognose che sono ancora ferite aperte per la Repubblica. Dobbiamo ricordarlo: l'affare della Locride, le tangenti per l'acquisto di aerei militari. Quelle erano vergogne.

Questa è la prima volta che un Ministro e un Governo - si può condividere o no - possono legittimamente venire nell'Aula del Parlamento

ma è e resta, com'è stato chiaramente indicato nelle memorie del Presidente del Consiglio, del vice Presidente Di Maio e del Ministro Toninelli, un'azione di Governo condivisa e portata avanti legittimamente. Non di immunità in questo caso si parla, dobbiamo essere chiari. Il MoVimento 5 Stelle non ha mai abdicato ai propri principi. *(Applausi

Io e i miei colleghi abbiamo votato perché andasse a processo la collega Paola Taverna, querelata, perché noi riteniamo che le immunità appartengano al passato e vadano superate. colleghi, quella che oggi affrontiamo è un'altra questione, che attiene al cuore della democrazia, alla possibilità di un Governo di compiere delle scelte. Queste scelte devono avere una valutazione. E la legge dice che la valutazione deve essere fatta in queste Aule, quando si tratta di un Questa è la rivendicazione che è nel DNA del Movimento, la restituzione della sovranità i cittadini, perché è in queste Aule che i cittadini esercitano la sovranità,

Non sto qui a ripetere ciò che altri, meglio di me, hanno già ripetuto. Non vi è dubbio che siamo in presenza di un'azione di Governo. Non vi è dubbio che questo bilanciamento di interessi nel caso di specie vi sia stato perché, a fronte di un interesse preminente, perseguito da anni dal Movimento, come quello di riportare l'Europa alle proprie responsabilità per il problema dei migranti, vi sia stato un sacrificio minimo, tollerabile in democrazia. Solo di questo noi dobbiamo parlare oggi in questa sede! Per questo motivo, annuncio, con orgoglio, che il MoVimento 5 Stelle, dopo avere condiviso 5 Stelle, dopo avere condiviso con i cittadini e i propri iscritti questa decisione, voterà convintamente affinché il Governo non debba rispondere di un'azione che è stata compiuta nell'interesse dello Stato e dei cittadini. *(I

i diritti umani rappresentano diritti inalienabili, che ogni essere umano possiede dalla nascita. Il riconoscimento della dignità specifica dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base di libertà, giustizia e pace nel mondo. I diritti umani sono iscritti e formano la base del diritto. Rappresentano forma superiore ad ogni altra norma. Detti diritti non possono essere compressi neanche un poco, salvo non siano un pericolo nel contingente di un bene giuridico costituzionale preminente dello Stato: dello Stato, che è di tutti, e non del Governo, che è di alcuni, come pericolosamente riportato nella relazione. Ebbene, i diritti umani dei membri della Diciotti sono stati compressi, in modo certamente reversibile, ma sono stati compressi. Diritti, tra l'altro, di soggetti fragili, tra cui minori, e in condizioni psicofisiche critiche. Questi diritti compressi devono essere comparati all'azione del Ministro, valutando se detta sottrazione sia valsa a tutelare un bene giuridico costituzionale preminente dello Stato. A mio giudizio, no. Aggiungo che è pericoloso, per ora e per il futuro, far passare il concetto che per far valere una finalità politica, un diritto, per quanto legittimo, verso altri, si possa far leva sui diritti di terzi, che nel caso specifico sono anche più deboli e in stato di disagio e fragilità.

Signor Presidente, il 5 aprile 2011 il Parlamento italiano votò che Ruby era la nipote di Mubarak e io mi chiesi spesso come fosse possibile negare l'evidenza per salvare la poltrona di qualche amico e mi ero detta che col MoVimento 5 Stelle questo non sarebbe mai più accaduto. Il vice *premier* Salvini ha detto una frase che mi è piaciuta: «a me dire le bugie viene poco e viene male». Anche a me dire le bugie viene poco e viene male, perché sono cresciuta nel MoVimento 5 Stelle con l'onestà come faro. Qui non c'era un interesse prevalente dello Stato, non c'era un interesse costituzionalmente rilevante a fermare 177 persone su una nave. C'era un interesse propagandistico; c'era un interesse politico con la «p» minuscola. Ho dato fiducia al Governo perché risolvesse il problema dei migranti e sono sicura che lo può fare con politiche intelligenti, lungimiranti e a lungo termine, ma non facendo questi giochetti.

verso quelle Forze dell'ordine che ha menzionato: le ragazze, i ragazzi, le mamme e i papà che ogni mattina mettono la divisa e scendono in strada a difendere la sicurezza nazionale, senza scorta e

Voglio ringraziare però i miei colleghi del Gruppo parlamentare e il capogruppo Patuanelli, che è sempre stato una persona aperta al dialogo, al confronto e alla trasparenza. Voglio ringraziare i miei colleghi con cui continuo ad avere un percorso insieme perché sono sicura che tutti loro in coscienza, qualunque cosa voteranno, lo faranno per tutelare il MoVimento 5 Stelle. E io, a differenza del ministro Salvini, affronterò un processo per questa mia scelta consapevole e coerente, perché sarò deferita ai probiviri, come giustamente vuole il codice del MoVimento 5 Stelle. Questo processo però io lo affronterò con la testa alta e la schiena dritta e avrei preferito affrontare un processo vero piuttosto che correre il pericolo di vedermi allontanata dalla magnifica comunità 5 Stelle. Solo una cosa posso dire

dunque alla votazione. Ricordo che la proposta della Giunta, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento, si intenderà respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 161 voti. Ricordo altresì che il risultato non verrà proclamato immediatamente. I senatori che non abbiano partecipato al voto potranno successivamente recarsi al banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali custoditi. Tale facoltà potrà essere esercitata fino alla chiusura delle operazioni di voto prevista per le ore 19. Concluse le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio e alla proclamazione del risultato. Ai sensi dell'articolo 135*-bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*. I senatori favorevoli alla proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere voteranno sì. I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro chiusa la votazione nominale con scrutinio simultaneo. Sospendo quindi la seduta, che riprenderà alle ore 17,30 per il sindacato ispettivo. Chiedo ai senatori Segretari di essere cortesemente presenti in Aula per raccogliere i voti fino alla ripresa della seduta.

economico*. Signor Presidente, in via preliminare all'illustrazione della risposta al presente atto di sindacato ispettivo vorrei innanzitutto evidenziare il lavoro svolto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, nel rispetto della tempistica programmata, sta garantendo la ricezione di tutte le domande dirette all'erogazione delle misure principali di questo Governo: il reddito di cittadinanza e quota 100. Il decreto-legge sul reddito di cittadinanza e quota 100 rappresenta, infatti, non solo un'importantissima misura di sostegno al reddito, che restituirà dignità a tutte quelle persone che oggi vivono intollerabili situazioni di povertà, ma anche quell'indispensabile investimento nelle politiche attive del lavoro, che nessuno dei precedenti Governi In questa prospettiva è chiaro a tutti che, per far fronte a queste nuove competenze, l'INPS ha avuto la necessità di adeguare il proprio assetto in modo da garantire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in modo rispondente a principi di efficienza ed efficacia che guidano l'azione pubblica. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, quindi, la riorganizzazione innovativa dell'area medico-legale dell'Istituto di previdenza appare finalizzata ad aumentare l'efficienza delle attività che ad esso fanno capo. L'INPS ha reso noto che detta riorganizzazione è fondata su criteri oggettivi che tengono conto sia del dato della popolazione residente, sia delle peculiarità legate ai carichi lavorativi. Il modello di presidio mira ad assicurare una copertura completa delle esigenze dell'intera platea di riferimento in campo previdenziale e assistenziale. L'accentramento delle attività medico legali, operato da tale modello organizzativo consente allo stato attuale una migliore ripartizione dei carichi di lavoro attribuiti ai singoli medici, nonché una migliore gestione degli aspetti organizzativi. Favorisce, inoltre, una migliore omogeneità valutativa garantendo maggiore trasparenza ed equità, a garanzia anche della correttezza, della collegialità e della legalità dell'azione accertativa. L'assetto descritto non esclude affatto, d'altra parte, la possibilità che per far fronte a specifiche necessità dei cittadini, vengano effettuati accessi domiciliari, ricorrendone i presupposti di legge e/o di opportunità. È chiaro che questa logica di adeguamento dell'assetto periferico dell'Istituto non dovrà mai tradursi in un disservizio per il cittadino e, pertanto, dal canto suo, il Ministero del lavoro

Governo, ringrazio il Vice Ministro e mi ritengo soddisfatto della risposta. Possiamo constatare, infatti, il fattivo impegno da parte del Ministero del lavoro nel porre la massima attenzione per evitare disservizi alla cittadinanza, a fronte degli adeguamenti periferici dell'Istituto. Concordo, quindi, pienamente con la linea del Ministero quando afferma che, all'aumento dell'efficienza dell'apparato organizzativo, debba corrispondere sempre una puntuale erogazione del servizio

con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che il Ministero dell'ambiente ha diretta competenza in materia di incendi per i piani antincendi boschivi delle aree protette statali, ossia i parchi nazionali e le riserve naturali statali, in attuazione dell'articolo 8, 2, della legge n. 353 del 2000, col supporto degli enti gestori di tali aree protette, che curano in modo particolare la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi. Spetta, invece, alle Regioni la diretta competenza sul resto del territorio per la programmazione e la pianificazione AIB e la lotta attiva anche all'interno delle suddette aree protette statali. Proprio al fine di realizzare iniziative di prevenzione volte a dare attuazione alle disposizioni della legge poc'anzi richiamata, il 9 luglio 2018 il Ministero dell'ambiente, l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno siglato un apposito protocollo d'intesa volto a definire le attività antincendi boschivi nelle aree protette statali, per poter contrastare al meglio il problema degli incendi boschivi in tali ambiti territoriali. Per quanto concerne, più nello specifico, le azioni antincendio nel territorio della Regione Puglia, la stessa ha fatto presente di aver adottato diverse iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Tra queste, ricoprono particolare rilevanza regionale n. 266 del 30 aprile 2018, recante «Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2018», che integra le norme generali di comportamento per contrastare gli incendi boschivi al fine di tutelare l'incolumità pubblica e il patrimonio forestale sul territorio regionale; nonché il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2018-2020, regionale n. 585 del 10 aprile 2018, che costituisce anche il presupposto per la elaborazione di ulteriori strumenti di programmazione degli interventi a tutela del patrimonio boschivo. Per quanto attiene le misure poste a tutela della Riserva naturale statale Le Cesine, si segnala che l'ente gestore (WWF) ha provveduto a predisporre il piano pluriennale AIB (2017-2021). Il suddetto piano prevede interventi selvicolturali per ridurre il potenziale innesco

tecnica dei Ministero dell'ambiente, sono stati acquisiti i pareri dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco ed è stata richiesta l'intesa alla Regione Puglia per l'inserimento del predetto piano AIB dell'area protetta nel piano AIB regionale. A ciò si aggiungano le iniziative già adottate dalla Regione Puglia per mitigare il rischio incendio nella suddetta Riserva, tra cui rientrano interventi di prevenzione attraverso l'istallazione di sensori per il superamento dei valori di ozono e anidride carbonica, finalizzali all'allertamento degli incendi mediante un progetto europeo, finanziato tramite la programmazione interregionale 2007-2013 e presentato dall'università di Lecce, con il coinvolgimento della sezione della Protezione civile regionale come *stakeholder*. La Regione ha rappresentato, inoltre, di avere in programma la realizzazione di un sistema di avvistamento a tutela della riserva. Sempre sulla base di quanto riferito dall'amministrazione regionale, con particolare riguardo alla lotta attiva agli incendi boschivi, la stessa ha provveduto a potenziare la capacità di contrasto sul territorio della provincia di Lecce, anche mediante la realizzazione di un campo operativo AIB di volontariato, gemellato con altre Regioni, presso il Comune di Campi Salentina. Inoltre, per sensibilizzare e informare la popolazione sul rischio incendi boschivi, ha programmato alcune giornate informative nei mesi di maggio e giugno 2018 e ha coinvolto le prefetture, le Forze dell'ordine, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Capitanerie di porto, i Comuni, gli enti gestori di servizi essenziali, gli enti gestori delle aree protette statali e regionali, le sezioni regionali competenti sulla materia e i coordinamenti provinciali del volontariato regionale di protezione civile. I sindaci coinvolti hanno provveduto a emanare apposite ordinanze, al fine di informare la cittadinanza. Nell'ambito delle predette attività di informazione, la Regione Puglia pubblica giornalmente sul proprio sito istituzionale il bollettino nazionale e regionale di previsione incendi. Per quanto concerne, infine, gli aspetti relativi alla qualità dell'aria in seguito all'incendio verificatosi nella riserva lo scorso mese di settembre, secondo quanto riferito dall'ARPA, i dati derivanti dalle attività ordinarie di monitoraggio non hanno mostrato superamenti dei limiti ambientali previsti dalla normativa di riferimento, di riferimento, né alcun incremento significativo delle concentrazioni degli inquinanti rilevati. L'ARPA ha comunque precisato che nelle immediate vicinanze dell'area dell'incendio non sono presenti stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria. Ad ogni modo, si aggiunga che l'Agenzia svolge il monitoraggio periodico delle acque, dei sedimenti e degli elementi di qualità biologici nell'area palustre che si trova all'interno dell'area interessata all'incendio. Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto e provvederà per il futuro alle attività e alle valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione e continuerà a monitorare l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di valutare possibili revisioni

Signor Presidente, se non ci fosse stato l'ultimo inciso dell'onorevole Sottosegretario, mi sarei dichiarato assolutamente insoddisfatto

È vero che la legge n. 353 del 2000 individua nelle Regioni gli organismi territorialmente competenti a verificare, controllare e programmare tutte queste attività, ma c'è quanto disposto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 che credo imponga al Ministero un' attività di coordinamento. Non ha una responsabilità diretta nella prevenzione e nell'attività necessaria alla prevenzione, ma sicuramente una responsabilità di coordinamento, di controllo e di stimolo degli organismi preposti. È evidente che se le Regioni non ottemperano a quanto la legge prevede, il Ministero può e deve intervenire per sollecitarle. Questo è il primo appunto che che ritengo di dover rappresentare all'esponente del Governo. Poi vi è un'altro aspetto. Non basta l'elencazione di tutte quelle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione degli incendi che sono previste dalla legge e che, quindi, devono essere fatte; noi ci aspettavamo dal Governo una risposta sull'effettiva attuazione e sul risultato raggiunto, perché molte volte l'attività di sensibilizzazione è un atto burocratico. Volevamo sapere se questo atto burocratico poi si fosse trasformato in una reale in una reale attività di sensibilizzazione e quali risultati si fossero raggiunti. Prendiamo atto con soddisfazione che, evidentemente, ci voleva questo incendio, che ha distrutto 50 ettari di macchia mediterranea,

con riferimento alle questioni poste, si ritiene opportuno evidenziare, in via preliminare, che il rilascio delle autorizzazioni agli impianti e la pronuncia dei pareri in merito a istanze presentate per la loro realizzazione sono di esclusiva competenza regionale e degli enti locali La Regione, nel rilasciare le autorizzazioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, tiene conto dei fabbisogni impiantistici e degli obiettivi contenuti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. A tal proposito, si precisa che, nel caso di specie, la Regione Sicilia è impegnata nell'adozione di un nuovo Piano di gestione dei rifiuti conforme al diritto europeo, che le permetta di raggiungere gli obiettivi nazionali di raccolta differenziata e di privilegiare le operazioni di gestione dei rifiuti poste ai livelli più alti della gerarchia. Il Piano è stato apprezzato dalla Giunta regionale nel mese di dicembre scorso ed è in corso la procedura di VAS regionale propedeutica alla sua approvazione Per quanto attiene, più nello specifico, alla realizzazione della piattaforma in argomento, il Comune di Centuripe ha fatto presente che la proposta presentata dalla Oikos SpA è stata inoltrata lo scorso settembre 2018, per il parere di competenza, agli enti preposti della Provincia di Enna, ossia l'azienda sanitaria provinciale (ASP), l'ufficio del genio civile e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. Con nota del 15 ottobre 2018 l'Azienda sanitaria provinciale ha ritenuto che si dovesse preliminarmente acquisire il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) parte dell'ARTA, nonché il giudizio preliminare da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Inoltre, sempre secondo l'ASP, la complessità progettuale dell'opera imponeva una valutazione in sede di Conferenza dei servizi. Il competente ufficio del genio civile di Enna ha richiesto, da parte sua, una modifica o integrazione della documentazione allegata alla proposta, al fine di poter esprimere il proprio parere a seguito di un compiuto esame. L'amministrazione comunale ha segnalato, inoltre, che è stata effettuata e trasmessa, previa richiesta della soprintendenza, la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico. All'esito dell'attività istruttoria finalizzata alla predetta verifica, la competente soprintendenza ai beni culturali e ambientali, con nota del 14 febbraio scorso, ha espresso il proprio parere negativo. Più in particolare, la predetta soprintendenza, considerato che l'area interessata dalla variante allo strumento urbanistico per la realizzazione del progetto comprende un'estesa porzione di territorio censita al catasto terreni del Comune di Centuripe e ricade in contrada Muglia, ha evidenziato che l'area è immediatamente contigua al sito d'interesse archeologico denominato Monte Pietraperciata,

Per queste ultime, ha precisato che il rinvenimento di reperti in dispersione sulla superficie delle stesse non esclude il rischio della presenza di reperti mobili o strutture nel sottosuolo. Il rischio archeologico basso è stato riconosciuto per una sola unità territoriale. Sempre secondo quanto evidenziato dalla soprintendenza nel proprio parere, l'esito positivo della verifica archeologica preliminare va confrontato con l'impatto che la realizzazione dell'impianto ha con il sottosuolo dell'area, dal momento che le opere previste comporteranno scavi, sbancamenti e un sostanziale sconvolgimento dell'attuale assetto pedologico e geomorfologico della porzione di territorio in oggetto. A tal proposito, la soprintendenza ha evidenziato, inoltre, che i terreni individuati per la costruzione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti sono compresi in una delle aree più dense di rinvenimenti archeologici della Sicilia centro-orientale, oltre che in uno dei comprensori paesaggistici isolani più integri e incontaminati dal punto di vista naturalistico. La soprintendenza ha concluso, quindi, ritenendo che la variante urbanistica proposta determinerebbe il cambiamento della destinazione rurale a cui l'area è vocata fin dall'antichità e che, stante il forte impatto ambientale delle opere in questione con le componenti naturali del sito, si finirebbe con l'arrecare grave pregiudizio alle valenze paesaggistiche dell'area soggetta a tutela. Sulla base di tali considerazioni, la soprintendenza ha pertanto espresso il proprio diniego alla proposta di variante allo strumento urbanistico avanzata dal Comune in ordine alla proposta di realizzazione della piattaforma. Alla luce delle informazioni esposte, si rappresenta che il Ministero continuerà comunque a monitorare la situazione e a tenersi informato mediante i soggetti territoriali competenti, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla vicenda.

vorrei esprimere in questa sede l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti in questa fase del procedimento autorizzativo rilascino, come ha fatto la soprintendenza di Enna, pareri preliminari che tengano conto delle caratteristiche e delle vocazioni proprie di quella porzione di territorio della Provincia di Enna di cui stiamo trattando. La cosiddetta piattaforma integrata di gestione e valorizzazione dei rifiuti che si intende realizzare in agro di Centuripe, a ridosso dell'abitato di Catenanuova, infatti, si configura come la più grande discarica mai realizzata in Sicilia. un impianto per la cui realizzazione sono già stati acquistati dalla società proponente circa 300 ettari di terra a vocazione fortemente agricola in un'area la cui produzione agroalimentare vedrebbe, inevitabilmente, compromessa la propria reputazione. Immaginate l'impatto che la presenza di una discarica di tali proporzioni avrebbe sulla salute della popolazione locale, che già adesso teme la prospettiva di vedere concentrati dietro casa un quarto di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Sicilia. Nei mesi scorsi migliaia di liberi cittadini, supportati da associazioni ambientaliste e culturali, hanno più volte manifestato in piazza per dire no alla realizzazione di quella discarica, spaventati dalla prospettiva certa di degrado del loro territorio, con grave danno per l'economia locale. Non riuscirò mai a comprendere l'atteggiamento di alcuni politici locali che affermano, con enfasi, di amare il proprio paese, ma anziché rilanciarlo attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, agroalimentare del territorio, cedono volontariamente alla proposta di realizzazione di una megadiscarica in grado di ricevere 1.000 tonnellate di rifiuti al giorno. Pochi giorni fa, ha avuto apparente conclusione la triste proposta di realizzazione di un'altra discarica, in questo caso per rifiuti speciali e pericolosi, da realizzarsi nei pressi di Agira, antico e orgoglioso centro nell'ennese, in un contesto ambientale e agricolo di comprovato pregio. Mi auguro che tale diniego sia definitivo e che in futuro non vengano concesse ulteriori autorizzazioni, anche quando limitate, ad esempio, ai soli manufatti in cemento-amianto: contrastare il multiforme ingegno di chi attenta all'ambiente con la malcelata connivenza di certi politici richiede, infatti, la massima attenzione. Considerato che la Regione Sicilia sta elaborando, come detto, un nuovo piano di gestione dei rifiuti, invito il Governo regionale siciliano ad affrontare il tema della gestione dei rifiuti in modo responsabile, senza permettere il saccheggio di un territorio ancora integro. È necessario - e mi piace ribadirlo in questa sede - puntare alla drastica riduzione dei rifiuti con politiche basate su prevenzione della produzione degli stessi, riutilizzo degli oggetti e riciclo dei materiali. Per far questo, bisogna realizzare impianti che consentano di chiudere il ciclo dei rifiuti, anche organici, differenziandoli in maniera sana ed efficiente, dando piena attuazione al principio dell'economia circolare. La Sicilia ha bisogno di tali impianti per archiviare la stagione delle discariche di vecchia concezione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, come detto, siamo nelle fasi preliminare di quello che ritengo un vero e proprio scempio, privo di senso, a danno di un territorio e della salute dei suoi abitanti: da rappresentante di quello stesso territorio mi opporrò con tutte le mie forze e nei limiti delle mie capacità, confortato anche dagli elementi acquisiti oggi, in quest'Aula.

ed alle ricadute negative che ne derivano sull'attuazione organica degli interventi atti ad attribuire alla pena il suo valore rieducativo, costituzionalmente garantito dall'articolo 27 della Costituzione. Si richiama, in particolare, la situazione della casa circondariale Gazzi di Messina, in cui per 272 detenuti vi sarebbero solo due funzionari giuridico-pedagogici, uno dei quali in congedo parentale saltuario, nonché la situazione della casa circondariale Sant'Anna di Modena dove, a fronte dei 484 detenuti, vi sarebbero solo cinque funzionari giuridico-pedagogici, due dei quali in distacco temporaneo ad altre strutture. Gli interroganti chiedono quindi di sapere se il Ministro interrogato non intenda avvalersi di ulteriori risorse nell'ambito giuridico-pedagogico, affinché si ponga rimedio alla problematica descritta. Va considerato in premessa che le dotazioni organiche complessive dell'amministrazione penitenziaria hanno subito un notevole ridimensionamento per effetto degli interventi di riduzione sugli assetti organizzativi previsti dalle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica.

mentre presso la casa circondariale di Modena non si evidenzia alcuna carenza al riguardo. Va altresì debitamente rimarcato che, a livello nazionale, il richiamato tasso di scopertura è destinato ad essere pressoché dimezzato in tempi brevi, in quanto è in fase di definizione la procedura finalizzata all'immediata assunzione di 37 unità

il trasferimento a domanda del personale dell'amministrazione penitenziaria inquadrato nel profilo professionale di funzionario giuridico-pedagogico, area terza, per la copertura di 39 posti complessivi, e che tra le sedi messe a concorso figurano proprio la casa circondariale di Modena e quella di Messina, entrambe per la copertura di un posto. Per completezza informativa, si evidenzia che con successivo provvedimento dello scorso mese di febbraio, si sono riaperti i termini del suddetto interpello essendo stati messi a concorso altri tre posti in altre sedi.

Prendo atto che il Ministero della giustizia si stia adoperando al fine di potenziare l'operato dei funzionari giuridico-pedagogici, aumentando la loro presenza all'interno degli istituti di pena. Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, il ruolo fondamentale rieducativo che la nostra Costituzione attribuisce alla pena detentiva: il detenuto deve essere messo nella condizione di poter formare e consolidare le proprie attitudini sociali e civili attraverso un percorso complesso, che non può e non deve prescindere dall'impegno e dalla competenza di personale qualificato. Competenza che nel nostro sistema penitenziario è rappresentata anche dai funzionari giuridico-pedagogici. È nell'ottica di quanto sopra esposto che apprendo con soddisfazione l'intenzione del Ministero della giustizia di dimezzare in tempi brevi il *deficit* di personale afferente all'area trattamentale mediante l'assunzione di nuovo personale. Nel caso specifico, gli interventi di ampliamento dell'organico previsto per le case circondariali Gazzi di Messina e Sant'Anna di Modena costituiscono un primo passo tangibile verso l'implementazione di una gestione virtuosa degli istituti di pena che nel nostro Paese è da sempre oggetto di gravi criticità. L'apprendere che le difficoltà del sistema carcerario italiano costituiscono una delle priorità del Ministero della giustizia ci permette di guardare con maggior fiducia al futuro di questo importante e delicato aspetto della sfera sociale del nostro Paese. *(Applausi

di affollamento pari al 105,37 per cento, come tale inferiore sia rispetto alla media nazionale, che si attesta sul 124,14 per cento, sia rispetto alla media regionale che si attesta sul 125,15 per cento. Per quel che attiene alla dotazione organica, occorre prendere le mosse dalla premessa di fondo per cui la riduzione la riduzione complessiva degli organici operata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, la cosiddetta legge Madia, e rivista dal decreto legislativo n. 95 del 2017, ha rimodulato la dotazione organica complessiva del Corpo, passata da 44.610 a 41.202 unità. La dotazione complessiva su base nazionale, alla data del 6 dicembre 2018, è rappresentata da 36.688 unità, con un tasso di scopertura dell'11 Presso la casa di reclusione di Asti risultano effettivamente presenti un totale di 168 unità rispetto ad una previsione organica pari a 186 unità, rilevandosi una percentuale di scopertura complessiva pari al 9,7 per cento, inferiore alla media nazionale. Nel ruolo degli agenti/assistenti presso l'istituto in esame non si registra alcuna carenza, bensì un esubero

di reclusione di Asti, tramite mobilità ordinaria dell'anno 2018, definita nel mese di settembre, è stata oggetto di un incremento di quattro unità maschili appartenenti alla qualifica degli agenti/assistenti. Inoltre, è prevista l'immissione in ruolo di 976 allievi vice ispettori che hanno frequentato il corso di formazione appena concluso. Quanto, invece, al ruolo dei sovrintendenti, sono tuttora in corso le procedure per il concorso interno a complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile del Corpo. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019/2012

circolare 9 ottobre 2018 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indirizzata a tutte le articolazioni centrali (direzioni generali) e territoriali (provveditorati regionali

Nello specifico, è stata dettagliata una mirata applicazione della normativa stabilita dall'articolo 42 della legge n. 354 del 1975, nella parte relativa ai trasferimenti per gravi motivi di sicurezza. Parimenti funzionale allo scopo è apparso il richiamo all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, nella parte in cui è prevista l'assegnazione, in via cautelare, a particolari

e non credo che solo una iniezione di polizia penitenziaria, pur sempre lodevole e ben accetta,

finestra") sul riordino della normativa concernente i servizi pubblici e gli adempimenti amministrativi di Province e Città metropolitane. Signor Presidente, signori senatori, il tavolo tecnico-politico previsto dal decreto legge n. 91 del 25 luglio 2018, si è insediato nella seduta della Conferenza Stato-Città del 20 dicembre scorso. I relativi lavori stanno proseguendo con continuità e fattività, in un clima di collaborazione e di proficuo confronto tra la componente governativa e quella delle autonomie locali, rappresentate da ANCI e da UPI, e sono finalizzati - com'è noto - alla redazione di linee guida in vista,di una necessaria revisione e sistematizzazione della normativa sull'organizzazione e il funzionamento degli enti locali, spesso oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi disarmonici e anche di dubbia efficacia. In particolare, con le linee guida si intende tracciare un percorso finalizzato alla revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni, alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto a quelli di piccole dimensioni. Dopo l'insediamento del tavolo si sono svolte diverse riunioni, nel corso delle quali sono stati esaminati ed approfonditi i contributi e le proposte avanzate dai rappresentanti delle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali. In prima battuta i lavori si sono focalizzati sulle modalità di realizzazione dell'associazionismo volontario dei Comuni in vista di un possibile e - aggiungo - necessario superamento dell'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali, in un'ottica di valorizzazione della loro autonomia, cosa ancor più cogente alla luce anche della recente sentenza della Corte costituzionale. Va considerato che l'esigenza di una riforma di tale ambito è legata principalmente al fatto che l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, imposto per legge ai piccoli Comuni, non ha prodotto i risultati attesi, dando vita sul territorio ad un associazionismo a macchia di leopardo, frutto anche dell'assenza di un'adeguata progettualità in materia, nonché di difficoltà di carattere procedurale. L'altro tema di cui il tavolo si è occupato e su cui ha focalizzato l'attenzione, che è in fase di avanzata definizione, è relativo alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, con specifico riferimento agli oneri a carico dei piccoli Comuni. In tale settore, occorre evidenziare come negli anni si siano moltiplicati, spesso in maniera incoerente con la capacità degli enti locali, adempimenti contabili e procedurali in misura tale da risultare particolarmente gravosi, rendendo sostanzialmente i Comuni stessi incapaci di assolvere ai medesimi. È emersa dunque la necessità di procedere ad un'opera di semplificazione degli adempimenti, in modo da consentire agli enti di governo del territorio di concentrarsi maggiormente sul versante dell'amministrazione attiva e della concreta cura degli interessi pubblici di riferimento. Aggiungo che nel corso dell'ultimo tavolo, svoltosi la scorsa settimana al Ministero dell'interno, abbiamo confezionato anche le linee guida sulla semplificazione degli oneri burocratici e amministrativi, addivenendo alla certezza su un principio chiaro ed evidente: non si può trattare nella stessa maniera soggetti oggettivamente differenti. I piccoli Comuni non possono avere le stesse regole dei grandi Comuni. Contestualmente, il tavolo tecnico-politico sta proseguendo il confronto sulle linee guida aventi ad oggetto la riforma delle Province e delle Città metropolitane. Il confronto sulle possibili modifiche ordinamentali e organizzative degli enti di governo di Area vasta è tuttora in corso e sono convinto che nelle prossime settimane le proposte avanzate dalle diverse parti potranno trovare un'utile sintesi. La funzione del tavolo è quella di indicare delle linee guida al Parlamento e al Governo. al Governo. Le linee guida saranno identificate anche eventualmente fotografando la divergenza di opinioni, ma certamente superando un'*impasse* legata ad una operatività che gli enti locali hanno sostanzialmente perso. In conclusione, il lavoro che stiamo portando avanti con il massimo impegno e con buoni risultati di confronto, nel rispetto della stringente tempistica, potrà costituire un'utile piattaforma per le successive iniziative legislative che, sono sicuro, riusciranno a recuperare a migliore utilità il ruolo delle Province, restituire centralità ai Comuni e a fare - ci si augura - finalmente decollare le funzioni delle Città metropolitane in definitiva a rispondere con maggiore efficienza ed efficacia ai bisogni e alle esigenze delle comunità locali. Dobbiamo ricordarci che anche dall'attività delle Autonomie locali deriva una gran parte dell'operatività degli investimenti. I nostri Comuni sono a loro volta sempre impegnati nella progettazione, ma troppo spesso ci sono difficoltà operative: il codice degli appalti ha la sua funzione, ma anche l'organizzazione stessa dei rapporti tra gli enti. Penso agli enti di area vasta, ovvero le Province, che hanno sostanzialmente perso una capacità operativa nel corso degli ultimi anni, dopo la cosiddetta riforma Delrio, fino ad arrivare alla moltiplicazione e alla nascita di una pletora impressionante di ambiti ottimali. Penso agli ambiti per la metanizzazione e ad altre strutture organizzative che sono sorte alternativamente alle Province, che, in effetti, danno luogo ad una non operatività. Basti pensare che nel corso degli ultimi due anni non è stato fatto un solo bando per la metanizzazione: ciò corrisponde anche ad ingenti investimenti che non vengono più realizzati sul territorio, perdendo non solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche in termini di urbanizzazione e di qualificazione dei servizi al territorio. Su questo stiamo lavorando; l'obiettivo è quello di giungere, nelle prossime settimane, come già accennavo, a una sintesi. Dopodiché, dovremmo metterci a riscrivere il testo unico degli enti locali, in accordo con il Parlamento, e certamente relazionandoci con tutti gli enti territoriali di rappresentanza: Comuni, Province e autonomie locali.

mi sembra che si sia iniziato e stia proseguendo un buon lavoro. Prendo atto del fatto che, finalmente, si vorrebbe mettere fine a una delle riforme obiettivamente - lo abbiamo detto tutti

follia. Credo sia molto importante - semplicemente perché lo si recepisce dal punto di vista dell'interlocuzione locale - l'elemento temporale.

Aggiungo il fatto che forse bisognerebbe cominciare a guardare alle macroregioni.

ha subito riavviato i lavori per la rielaborazione dello schema di decreto FER finalizzato a incentivare le fonti rinnovabili, in conformità ai propri orientamenti politici in materia, segno della volontà di proseguire e rafforzare il sostegno al settore. Il citato schema è stato, dunque, concertato con il Ministero dell'ambiente e sono stati acquisiti i pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e della Conferenza unificata. A fine gennaio 2019 il testo è stato infine notificato alla Commissione europea per la verifica della sua conformità alle norme comunitarie e, segnatamente, alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (di cui alla comunicazione della Commissione europea n. 2014/C 200/01). È già iniziata, di conseguenza, l'interlocuzione con i servizi della Commissione europea che ha formulato dei chiarimenti cui i Ministeri interessati hanno lavorato, presentando le relative risposte in occasione della videoconferenza tenutasi il 14 marzo scorso. In quella sede, la Commissione ha anche chiesto di motivare in modo più articolato alcune scelte inserite nel decreto. Si conta di riscontrare al più presto tali istanze in modo da pervenire all'approvazione del regime in tempi rapidi, tenendo conto della circostanza che la Commissione ha sessanta giorni di tempo dalla notifica per dare il via libera allo schema di decreto, termine che tuttavia potrebbe iniziare a scorrere di nuovo nel caso di ulteriori richieste istruttorie, anche se per tali motivi il *timing* delle procedure per l'assegnazione degli incentivi inizierà nel 2019. far presente che il *budget* e i contingenti di potenza incentivati saranno sensibilmente aumentati rispetto all'originaria previsione. Le tecnologie oggetto del decreto notificato sono quelle più mature, con costi prevalentemente fissi, bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione (eolica *onshore*, solare fotovoltaica, idroelettrica e gas residuati dei processi di depurazione), mentre le fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovatività nel contesto nazionale, con costi fissi ancora elevati o tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di esercizio (eolica *offshore*, energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia, ivi inclusa la geotermia convenzionale) sono inserite in un altro decreto in corso di preparazione. A margine va ricordato che il Governo italiano, il 28 dicembre scorso, ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di Piano integrato per il clima

e alle opportunità economiche ed occupazionali per le famiglie e il sistema produttivo. Una delle novità contenute nel citato Piano, anche alla luce della direttiva RED UE/2018/2001, è rappresentata dal maggior coinvolgimento del cittadino (che assumerà un ruolo centrale anche nella veste di *prosumer*) e delle imprese, in particolare di quelle medie e piccole. Vorrei infine evidenziare che che il decreto che si è notificato, sebbene sia da collocare tra le misure per il raggiungimento degli obiettivi al 2020, rappresenta in ogni caso l'occasione per sperimentare alcuni strumenti di sostegno innovativi, quali ad esempio la promozione dell'autoconsumo, l'utilizzo del fotovoltaico in sostituzione di coperture in amianto e i PPA (*power purchase agreement* o contratti a lungo termine), che potranno essere implementati anche in vista degli obiettivi al 2030, quale integrazione o alternativa ai regimi di sostegno tradizionali.

auspichiamo una celere emanazione del provvedimento, visto che i settori interessati sono da tempo in attesa e ci auguriamo che le richieste della Conferenza unificata tra Stato, Regioni e Comuni e della Commissione europea sull'incentivazione del geotermoelettrico e del mini e medio idroelettrico siano recepite nel testo finale.

Signor Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, intervengo perché il 1° marzo 2019 mi sono recato in visita presso il Comando militare esercito (CME) dove ho avuto modo di conoscere sia il livello d'integrazione sul territorio del Comando molisano, unico ente dell'Esercito presente in Regione, sia la professionalità e la determinazione di tutto il personale, che da sempre rappresenta un sicuro punto di riferimento per l'intera comunità molisana. La conoscenza derivatami a seguito della visita mi ha fornito la matura consapevolezza nell'affermare che il previsto provvedimento di soppressione del CME Molise, derivante dal decreto legislativo n. 7 del 28 gennaio 2014, non potrà e non dovrà essere eseguito. Il decreto legislativo n. 7 menzionato prende ispirazione da una logica di natura aziendale, per cui un provvedimento di soppressione di un ente dovrebbe dipendere dalla scarsa produttività o dagli eccessivi costi di esercizio. Proprio questi due indicatori non trovano correlazione e applicazione al Comando molisano, perché, per quanto riguarda l'indice di produttività, l'ente è al di sopra di molti reparti insistenti in Regioni ben più popolose. Per quanto riguarda, invece, i costi di gestione, che ammontano a circa 60.000 euro l'anno, l'eventuale chiusura paradossalmente graverebbe sul bilancio dello Stato per diverse centinaia di migliaia di euro, in virtù della legge 29 marzo 2001, n. 86, che disciplina il trasferimento del personale militare. la ragione fondamentale per la quale la paventata chiusura del Comando militare esercito Molise non potrà essere eseguita è perché, per la prima volta nella storia unitaria italiana, una Regione non avrebbe più alcun presidio militare sul territorio (precedente, questo, unico e inaccettabile). Da ultimo, ma non meno importante, la sciagurata ipotesi di una soppressione aprirebbe la questione delle emergenze. A tal proposito, mi preme ricordare che il territorio molisano è considerato, così come la storia ci ha più volte insegnato, tra le zone a più alto rischio sismico d'Europa. Per tali ragioni, credo che i cittadini molisani non debbano ulteriormente veder depauperata la presenza di presidi dello Stato sul territorio. In conclusione, chiedo che il Ministero della difesa si adoperi per garantire il mantenimento del presidio sul territorio, auspicando anche, ove possibile, un ampliamento delle sue funzioni.

Presidente, colleghi, ho chiesto di intervenire in Aula per richiamare un fatto molto grave, ossia la manifestazione prevista per sabato prossimo, indetta da Forza Nuova per celebrare il centenario della nascita dei fasci italiani di combattimento, combattimento, autorizzata questa mattina nella città di Prato. Ci sarà tempo per capire le responsabilità dei vari livelli istituzionali in questa vicenda, ma voglio fare un ultimo appello al Governo, tramite la Presidenza del Senato, perché impedisca questa manifestazione. Ricordo che in Italia l'apologia del fascismo è reato, introdotto nel 1952 dalla cosiddetta legge Scelba allo scopo di attuare la XII disposizione transitoria della Costituzione che recita: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». La legge non punisce soltanto la riorganizzazione, ma anche tutti quei comportamenti che esaltano il fascismo. La norma sanziona chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Dopo diversi anni è intervenuta la cosiddetta legge Mancino a specificare ulteriormente quanto previsto dalla legge Scelba. La legge, approvata nel 1993, punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e l'esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Consentire un raduno di fascisti in una città come Prato, decorata con la medaglia d'argento al valor militare per la guerra di liberazione, in un contesto politico come quello attuale, che vede il clima sempre più surriscaldarsi, è una responsabilità grave di cui il Governo deve essere consapevole. Oltre 16.000 cittadini hanno firmato negli scorsi giorni un appello perché la manifestazione non si tenga. Il sindaco ha chiesto che venisse negata l'autorizzazione e così hanno fatto la Curia e molte associazioni libere e pacifiche che si ritroveranno a Prato per un presidio pacifista e antifascista, in contemporanea alla manifestazione di Forza Nuova. Ieri mattina la città di Prato si è svegliata con svastiche sui muri delle sedi dell'ANPI e del Partito Democratico, corredate dalla scritta: «Arriviamo». Cosa ancora deve succedere perché si capisca che questa manifestazione va fermata? Non lo so, ma è giusto che ognuno si assuma le responsabilità che gli competono. Per questo motivo ci tengo a lasciare agli atti questa mia dichiarazione nell'Aula del Senato, affinché dopo non si dica che nessuno l'aveva detto. **Saluto

di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola in quest'Aula per portare all'attenzione una problematica sentita da me e da molti e alla quale credo sia arrivato il momento di dare una risposta fattiva e concreta. Mi riferisco ai continui episodi di violenza nei confronti dei direttori di competizioni sportive. La situazione è grave e merita, a mio avviso, un intervento del legislatore volto a contrastare la spirale di violenza che tanto si allontana dai valori fondanti dello sport, quello sano da intendersi come palestra di vita per le giovani generazioni. Sono valori che abbiamo il dovere di tutelare e difendere. Tra le ultime vicende in ordine di tempo c'è l'aggressione a Tiziano - dico solo il nome - con calci e pugni al termine di uno spareggio di un campionato *under* 17.

che ha l'obiettivo di assegnare la competenza al tribunale ordinario in composizione monocratica del delitto di lesioni personali lievi e lievissime, di cui all'articolo 582 del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni di carattere sportivo. Sulle finalità del provvedimento ho riscontrato un'ampia condivisione da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione. Presidente, si entra nel campo con la paura che un proprio errore di valutazione, una semplice distrazione o semplicemente che una decisione non condivisa possano tradursi poi in violenza. A questo si è arrivati a causa di una sciagurata e deforme interpretazione dello spirito sportivo da parte di alcuni (fortunatamente si tratta Credo sia arrivato il momento di dire basta e di porre rimedio a una situazione che ormai è insostenibile per la classe arbitrale e per quanti hanno voglia di continuare a credere nei valori che poc'anzi richiamavo e di cui lo sport è portatore essenziale e primario. *(Applausi

spinse il Governo Renzi al disastro Etruria. Adesso la Corte di giustizia lo annulla». Volevo, quindi, richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del Governo su uno dei più gravi scandali riguardanti il risparmio degli italiani, tutelato dell'articolo 47 della Costituzione. hanno visto azzerati i loro risparmi da decisioni sciagurate e arbitrarie della Commissione europea con la direttiva BRRD, meglio conosciuta come *bail in*, un vero e proprio esproprio criminale del risparmio avallato dall'allora Governo, sulla cui paternità e approvazione ho visto scorrere in questi ultimi mesi abbondanti quanto beffarde lacrime di coccodrillo. in particolare, alla decisione della commissaria europea per la concorrenza Vestager, pochi giorni fa addirittura osannata pubblicamente nel corso di un'audizione in Senato, che bollò come aiuti di Stato il legittimo intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che nel 2015 effettuò il versamento di 265 milioni di euro alla Banca popolare di Bari a copertura delle perdite per l'acquisizione della Tercas imposta dalla Banca d'Italia. Quella decisione illegittima, contraria all'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, all'origine della risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, oltre ad aver bruciato i risparmi di 130.000 famiglie con l'anticipo del *bail in*, costò oltre 5 miliardi di euro solo per ripulire le quattro banche e comportò una valutazione delle sofferenze al 17,6 per cento del valore di riferimento, svilito Si tratta di decine di miliardi di euro diventati, per taluni banchieri e fondi avvoltoio, l'affare del secolo. Quella decisione scatenò un'altra catena di eventi sulle modalità dei successivi salvataggi bancari, sia per MPS che per altre banche. che per altre banche. Ci furono danni tangibili e quantificati dal presidente della Banca popolare di Bari, Marco Jacobini, in un miliardo di euro perso per la raccolta e danni reputazionali per i risparmiatori. Concludo dicendo che è sconvolgente lo scaricabarile della commissaria Vestager, che cerca di addossare la responsabilità su Bankitalia. Noi che non abbiamo mai fatto sconti a Bankitalia, auspicando che chiarisca e reagisca, cercheremo di presentare una mozione per chiedere al Governo di intervenire con la sacrosanta richiesta dei danni ad una Commissione europea che ha deliberatamente provocato la crisi bancaria in Italia, mettendo sul lastrico 300.000 famiglie.

ma poi non controlliamo ciò che realmente succede nella vita reale. Oggi, dalle mie parti, un senegalese con precedenti penali alla guida di un bus ha sequestrato 51 ragazzi, legandoli,

un gesto ignobile nei confronti di poveri ragazzi che stavano andando a scuola per svolgere le ore di ginnastica. Quei ragazzi potevano essere i nostri figli, i miei figli!

però la domanda che faccio e la riflessione che voglio condividere con voi è: come è possibile che nel 2019 una persona con precedenti penali possa guidare un bus pieno di bambini? Questo non riesco proprio a concepirlo intervento ringraziando i carabinieri di San Donato Milanese e di Segrate per l'ottimo intervento e per aver portato in salvo tutti i bambini.